Signor Presidente del Senato, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, il Consiglio europeo di domani e dopodomani ha diversi punti all'ordine del giorno il primo dei quali, primo almeno dal punto di vista dell'interesse generale, riguarda la discussione sul futuro dell'Unione.

perché credo siamo tutti consapevoli del fatto che nei prossimi quindici o sedici mesi, prima della conclusione di fatto della legislatura europea e dell'avvio della campagna per il rinnovo del Parlamento e delle istituzioni europee, esistono diverse opportunità per fare dei passi in avanti. Il quadro in cui tale discussione si colloca è tutto sommato favorevole. Abbiamo dei numeri all'economia europea, in particolare dell'eurozona, che sono complessivamente favorevoli (certo, se paragonati alla crisi degli anni precedenti); abbiamo un tasso di crescita dell'eurozona del 2,2 per cento, piuttosto stabile nelle sue previsioni; abbiamo di

e cioè le dinamiche che il voto - che ovviamente rispettiamo, essendo espressione democratica della volontà dei cittadini britannici - ha provocato, cioè un processo interno al Regno Unito che non pare caratterizzato, almeno non fino ad ora, da grandi successi, grandi risultati ed entusiasmanti conseguenze politiche ed economiche. Detta più semplicemente, in Europa abbiamo l'impressione che decisioni come quella presa dal Regno Unito di uscire dell'Unione europea non siano portatrici di conseguenze straordinariamente positive pur meritando, lo ripeto, tutto il nostro rispetto. Abbiamo avuto risultati elettorali certamente disomogenei, diversi tra loro in diversi Paesi europei ma che complessivamente confermano la forza e la solidità dell'impianto delle forze politiche e di Governo che per l'Europa sono impegnate. impegnate. In questo contesto favorevole può svilupparsi una opportunità, una possibilità positiva. Noi, per la verità, l'avevamo in parte già colta, se ricordate, qui a Roma nel marzo scorso, in quell'appuntamento tutt'altro che celebrativo per i sessant'anni dei Trattati in cui abbiamo avuto la netta sensazione che l'inverno dello scontento europeo si fosse in qualche modo, forse, sciolto nella nella bellezza della Roma di marzo, o per lo meno avevamo avuto l'impressione di una reazione a Brexit e alle difficoltà che erano state incontrate. Questo sarà il primo punto in discussione al Consiglio europeo: come approfittare di questa finestra di opportunità, come rispondere alle sollecitazioni che da Roma in avanti sono venute nelle forme più varie e ultimamente sono venute da alcuni discorsi importanti, il discorso del presidente Juncker sullo stato dell'Unione europea e il discorso del neoeletto Presidente francese alla Sorbona, discorsi che hanno cercato di dare una spinta nel senso della costruzione europea, anche accettando l'idea che sia possibile immaginare un livello diverso di integrazione tra i diversi Paesi senza cambiare e modificare i Trattati e utilizzando le regole esistenti.

Dobbiamo stare molto attenti a non passare da una situazione di tempesta perfetta, che sembrava attraversare l'Europa un anno e mezzo fa, caratterizzata da crisi economica, difficoltà e ad una condizione di occasioni mancate che, potrebbe caratterizzare l'Europa dei prossimi mesi, se non diamo alla discussione sul futuro la dimensione che merita dal punto di vista politico e operativo.

nella parte in cui si è sempre collocata nei decenni, cioè tra i Paesi che ritengono sia giusto spingere per un livello maggiore di integrazione europea. Questa è sempre stata la posizione del nostro Paese nei decenni e credo che ci siano tutte le condizioni per considerare la posizione a favore di un livello maggiore di integrazione europea come quella che va incontro ai nostri interessi nazionali. Su alcuni temi si faranno dei passi in avanti già domani e dopodomani: penso alle politiche europee di cooperazione rafforzata sulla difesa, su cui ci saranno dei nuovi piccoli passi in avanti; penso all'Europa digitale, argomento di cui si è molto parlato in Estonia e che vedrà nel Consiglio europeo di domani e dopodomani la decisione di esaminare esaminare le proposte della Commissione anche a proposito di una *web tax* europea per quanto riguarda i grandi giganti e le grandi piattaforme del *web*. prospettiva che non esclude e, anzi, in fondo fornisce un ombrello protettivo ad eventuali decisioni nazionali che comunque anticipino questa direzione. passi quindi si faranno e, tuttavia, dobbiamo essere consapevoli che siamo ancora lontani dal definire un programma di svolta per l'Unione europea per quello che riguarda le prospettive di un'Unione della crescita e del lavoro. Le proposte italiane di questi anni sono state relative ad un'Unione capace di proporre un meccanismo di assicurazione europea contro la disoccupazione in casi di *shock* asimmetrici nelle economie europee. Un'Unione capace di investire sui beni comuni europei, magari, in una prima fase, sottraendo gli investimenti sui beni comuni europei dal computo del *deficit* e del debito e, in un seconda fase, investendo sui beni comuni europei con risorse proprie. Di qui, tutto l'argomento del bilancio proprio dell'Unione europea, su cui molto si è lavorato a livello tecnico: ricordo la relazione svolta dal professor Monti e i tanti contributi che sono arrivati in questa direzione. Un'Unione che pensa ad un Fondo monetario europeo e ad un Ministro dell'economia europeo e naturalmente pensa a queste figure non come all'introduzione di un revisore dei conti europeo che va a prendere le misure degli scostamenti in questo o quel Paese discolo (magari meglio se mediterraneo), ma come un Fondo monetario europeo e un Ministro dell'economia europeo che siano in un rapporto politico con il Parlamento e abbiano un ruolo di promozione dell'Europa del lavoro e degli investimenti. Questa è la strada verso la quale dobbiamo andare. Non possiamo accettare l'idea che il dibattito sul futuro dell'Unione europea diventi una sorta di azione parallela, di cui si discute nei vertici, più o meno frequenti, e all'ombra della quale vengono avanti, magari sul piano tecnico, decisioni e impostazioni, che vanno in direzione completamente diversa. Se questo è il terreno di avanzamento dell'Unione europea, ciò deve tradursi in scelte politiche, economiche e di governo a livello europeo. Questa è la spinta dell'Italia e su questo credo che l'Italia debba presentarsi con il sostegno il più possibile unitario del Parlamento.

dall'Europa della crescita, degli investimenti, di un bilancio comune e, certamente, da un'Europa in grado di sviluppare politiche migratorie comuni.

che, da un lato, possiamo essere orgogliosi, come Italia, del fatto che in questi anni siamo stati un Paese all'avanguardia nel salvare vite umane nel Mediterraneo e questo lavoro e questo valore della nostra politica ci sono stati sempre riconosciuti a livello europeo.

in particolare negli ultimi mesi, sviluppando la propria iniziativa politica, a infliggere un colpo molto rilevante all'assoluto predominio dei trafficanti di esseri umani nei flussi migratori del Mediterraneo centrale. Questo è il risultato che possiamo rivendicare in sede europea: da un lato siamo il Paese impegnato a livello umanitario, che salva vite umane e dà il buon esempio nel Mediterraneo e, dall'altro, siamo il Paese che mostra che è possibile sconfiggere il traffico illegale di esseri umani e ridurre i flussi migratori. Onorevoli senatrici e senatori, non c'è un'altra strada per gestire la questione migratoria nei prossimi dieci, venti Chi si illude che ci possa essere un modo per cancellare improvvisamente dalle pagine della storia e della geografia i flussi migratori si sbaglia e illude i nostri concittadini. Una cosa certo, è possibile: andare verso una situazione gestita, in cui i flussi migratori irregolari vengono ridotti nel numero, controllati dal punto di vista della sicurezza e gradualmente trasformati in flussi regolari. Questa è la sfida che abbiamo davanti e noi ci presentiamo in Europa, forse mai forti come adesso, nel dire che l'Italia ha mostrato la strada e abbiamo bisogno che gli altri Paesi dell'Unione europea su questa strada si impegnino e ci diano una mano. Il calo che abbiamo avuto negli arrivi non è un numero da esibire per ragioni di consenso elettorale. È molto importante che si sia ridotto il numero degli arrivi irregolari gestiti dai trafficanti, che come sapete si è ridotto in modo molto significativo nel corso dell'anno, in modo particolare negli ultimi tre o quattro mesi, ma è molto importante perché questo calo consente una gestione ordinata dei flussi e consente gradualmente di spostare verso i Paesi di transito e verso i Paesi di origine il peso di tale fenomeno. Ma lo spostamento è possibile se è frutto di un investimento e di un impegno di tutti i Paesi europei. Non esiste una politica migratoria di successo in un Paese solo. Non esiste la possibilità di risolvere la questione soltanto da parte dell'Italia, per quanto l'Italia abbia fatto progressi, passi avanti e ottenuto successi.

uno o due Paesi europei. Vi è riluttanza nel mettere risorse per finanziare il lavoro che si sta facendo in Libia o in Niger per i rimpatri volontari e rendere umani e rispettosi dei diritti umani i campi dei rifugiati in Libia. È un lavoro insufficiente. Finalmente si stanno aprendo questi spazi. Potremmo addirittura arrivare, nelle prossime settimane, al risultato dell'apertura di un primo campo

L'OIM, l'Organizzazione internazionale per i migranti, che si occupa dei migranti non rifugiati, quest'anno arriverà forse a oltre 10.000 rimpatri volontari dalla Libia verso altri Paesi africani. Qui si intravede una soluzione strategica del fenomeno, non per cancellarlo, ma per renderlo gestibile, approfittare dei suoi aspetti positivi e ridurne l'impatto sociale negativo. Ma se l'Europa non si mobilita e se i singoli Paesi europei, al di là dell'impegno della Commissione e di un contributo che è venuto da Paesi come la Germania, non si muovono in questa direzione, rischiamo di rimanere sospesi in questo lavoro e fare dei passi avanti ma lasciarli lasciarli fragili e non arrivare alla conclusione che sarebbe necessaria. Quindi, chiederemo, nel vertice di domani e dopodomani, un impegno maggiore sul piano economico di tutti i Paesi membri e il presidente Tusk mi ha assicurato che sarà il primo a fare questo appello in apertura dei lavori. Chiederemo un impegno dei diversi Paesi a sostenere i risultati della politica italiana: non discorsi generici, ma risultati

la Spagna (anche se finora non ci sono numeri significativi in quella direzione), il peso dei grandi flussi che vengono dall'Africa o dal Medio Oriente verso il Mediterraneo. E non possiamo accettare che, mentre si è molto stretti nella collaborazione su tali politiche, si chiedano chiusure sempre più rigide per quanto riguarda i confini interni all'Unione europea. Onorevoli senatori, ho sentito qualcuno in Italia rallegrarsi per il successo di questa o quella formazione politica in qualche Paese europeo che fa del sigillare le frontiere contro l'Italia una sua grande bandiera. C'è poco da rallegrarsi

fieri né da incoraggiare. Dobbiamo incoraggiare l'impegno in Africa, in Libia, nella solidarietà con i Paesi di primo arrivo, non incoraggiare chi vuole sigillare le frontiere europee rendendo ancora più difficile la situazione dei Paesi in prima linea.

Sapete che nella discussione in Europa la trattativa con Londra è stata impostata individuando due diverse fasi di questo confronto. confronto. Una prima fase si affronta la questione economica, cioè i fondi che il Governo britannico deve restituire all'Unione europea nel momento in cui abbandona l'Unione. altresì la questione di un Paese europeo che confina direttamente con il Regno Unito, cioè l'Irlanda, ossia che cosa succede in quei delicatissimi confini all'interno dell'Irlanda nel momento in cui le due parti dell'Irlanda non fanno più parte entrambe dell'Unione europea. In terzo luogo, vi è la questione a cui noi italiani siamo forse, come Governo nazionale - anche se ovviamente ci interessa l'insieme più direttamente interessati: che cosa succede ai cittadini europei che vivono e risiedono nel Regno Unito. Noi abbiamo infatti centinaia di migliaia di italiani che vivono e risiedono nel Regno Unito e devono avere il messaggio, da Roma, dal Parlamento, dal Governo, che i loro diritti saranno difesi da parte nostra e che non accetteremo, sull'altare della Brexit, che vengano Il Governo britannico - anche ieri ho ricevuto una telefonata molto cortese del primo ministro May - preferirebbe che la discussione sull'assetto futuro dei rapporti tra Regno Unito e Unione europea cominciasse anche prima del previsto e quindi che la sequenza tra discussione sui tre *dossier* e discussione sui rapporti futuri fosse in qualche modo incrociata; in altre parole: «aiutateci cominciando a discutere subito dei rapporti futuri tra Gran Bretagna e Unione europea, senza chiederci di chiarire prima sui soldi, sui confini con l'Irlanda, sullo *status* dei cittadini». Penso che noi dobbiamo un atteggiamento amichevole nei confronti del Regno Unito, come l'abbiamo sempre avuto nella nostra storia, per motivi che ben conoscete, e che possiamo anche accettare l'idea che ai livelli tecnici si cominci a discutere degli assetti futuri. Ma, se nel prossimo Consiglio europeo di dicembre si vuole cominciare a discutere degli assetti futuri, bisognerà aver fatto, prima di questo, dei passi in avanti sostanziali nei tre *dossier* che ho citato prima, altrimenti sarà molto difficile cominciare la discussione sul futuro senza aver posto neanche le premesse dal punto di vista finanziario e di bilancio. Infine, onorevoli senatrici e senatori, dentro il discorso della Brexit c'è anche, come sapete, la discussione sul destino delle due agenzie europee europee importanti che hanno sede a Londra: l'Agenzia delle banche e quella del farmaco. Non sarà una decisione che si prenderà nel Consiglio europeo, ma può darsi che l'argomento venga tuttavia sfiorato

dall'Agenzia europea del farmaco e dalla Commissione europea nei loro *assessment*, nelle loro valutazioni - che la candidatura italiana della città di Milano

Con tutto il rispetto (che non è formale, perché io mi rendo perfettamente conto di questo problema e di questa esigenza) che si deve al principio dell'equilibrio geografico nei confronti di Paesi che, essendo entrati più tardi nell'Unione europea, non hanno ancora il privilegio e la possibilità di ospitare delle agenzie europee, con tutto il rispetto per questo principio, io ritengo che esso non possa andare a discapito della qualità e della funzionalità di una agenzia così importante per la salute,

non nel caso di un'agenzia che ha bisogno, dal primo giorno dopo il suo trasferimento, di funzionare a pieno regime. Di nuovo, viene qui alla luce uno dei nodi della discussione sul futuro dell'Europa. L'Italia non ha mai avuto un atteggiamento sprezzante verso i Paesi di nuovo ingresso. Anzi: il loro ingresso sanciva una grande stagione di libertà in Europa. Il Presidente della Commissione europea, nel periodo in cui questo ingresso vi fu, era del resto un italiano. Quindi, ci mancherebbe altro che noi fossimo contrari a riconoscere l'importanza e il ruolo di questi Paesi di nuovo ingresso. Dobbiamo, però, avere in mente quali sono gli obiettivi del progetto europeo; la loro qualità, la loro ambizione. Essere uniti a resta un requisito fondamentale. Ma questa unità non può essere un peso rispetto all'ambizione e al futuro del progetto europeo. Vale per le agenzie e vale per l'orizzonte europeo comune che ci lega. Al riguardo io credo che il Governo possa contare su un consenso vasto in Parlamento, che rende più forte la sua posizione al tavolo di Bruxelles. *(Applausi

Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, condivido pienamente le sue valutazioni e gli orientamenti politici che ha espresso in ordine sia ai problemi dell'agenda europea sia al contributo che l'Italia può e deve dare in questa fase nell'interesse dell'Europa ma anche proprio. Per i motivi che lei ha indicato i prossimi quindici o sedici mesi possono rivelarsi decisivi. Ne aggiungerei un altro di motivo, al quale ella comunque ha fatto allusione: nel maggio prossimo la Commissione europea presenterà la proposta di quadro finanziario pluriennale per i sette anni che inizieranno nel 2021. Quindi, si arriva al 2027. Se ne parla ancora poco, ma come lei sa, signor Presidente, si stanno scaldando i motori. Quali vogliamo siano i compiti dell'Unione? Che cosa deve fare più o meglio di oggi? Che cosa deve fare meno di oggi? Quanto dovrà destinare, ad esempio, a una politica della difesa comune? Quanto alla politica agricola? Come dovrà finanziarsi? Dovrà o no avere risorse proprie? Ripeto che ci sarà una proposta della Commissione nel maggio 2018 e l'obiettivo della Commissione è di raggiungere una decisione con Consiglio e Parlamento prima delle elezioni europee del maggio 2019. Questa sarà una decisione che plasmerà l'Unione e gli Stati membri, dunque anche l'Italia, fino a dieci anni da oggi. come lei ha detto, ai tavoli di queste decisioni, così come di quelle su crescita e occupazione, il Paese deve presentarsi, se possibile, unito e comunque forte nelle proprie determinazioni. ultimi anni, con una continuità di impegno che lei ha sottolineato, il nostro Paese ha rimediato a diverse delle proprie debolezze e vulnerabilità e rafforzato diversi suoi punti di forza. Vi è ancora, tuttavia, una complessiva percezione di scarsa solidità del nostro sistema, di non piena affidabilità rispetto agli impegni presi. Questo vale presso gli osservatori politici e, tutt'ora, nei mercati. vi sembra normale che oggi lo *spread* nei confronti della Germania sia di 163 punti per l'Italia e di 120 per la Spagna? Questo è un differenziale che paghiamo tutti: Stato, imprese e famiglie che ricorrono a mutui. È vero che il debito pubblico dell'Italia è molto superiore a quello della Spagna, ma la Spagna è un Paese che ha rischiato - e forse rischia ancora - la rottura della Nazione. Allora, cosa possiamo fare - Governo, Parlamento, partiti e società civile - per convincere la famiglia europea, nel nostro interesse e non tanto nel loro, che l'Italia è una componente solida, convinta, certo assertiva, non passiva e remissiva, di un'Europa che tutti vogliamo rafforzare? Cosa possiamo fare? Vorrei esprimere un auspicio in quest'Assemblea. Ho l'impressione che tra noi, nell'arena della politica interna, si registrino, in realtà, sul grande tema dell'Europa e delle sue diverse articolazioni, divergenze un po' minori rispetto a qualche tempo fa e a quelle che appaiono spesso moltiplicate ed esagerate all'estero. Voi sapete, per la mia storia personale, che non ho né avversioni, né appartenenze e che guardo con rispetto alle diverse opposizioni, così come alle diverse componenti della maggioranza. Ebbene, mi sono chiesto che cosa potrebbero fare in questo momento le opposizioni e la maggioranza per rendere più riconosciuta la presenza dell'Italia, oltre alla grande azione che sta svolgendo il Governo con il Presidente del Consiglio, in Europa.

che in passato si erano marcate per una distinta posizione ultradialettica nei confronti dell'Europa, espressioni più riflessive e pragmatiche. C'è un modo per mostrare anche all'estero che non è più vero che, in caso di determinati esiti elettorali, dall'indomani l'Italia uscirebbe dall'euro e dall'Unione europea? Mi sforzo di spiegarlo quando vengo interrogato e spero che sia vero, ma forse si può fare qualcosa di più per non far pagare a tutto il nostro Paese una percezione che forse non è più molto attuale e corretta all'estero. adesso rivolgermi simmetricamente ai senatori del Partito Democratico, partito che ha avuto un ruolo importante in tutto il percorso dell'Italia fino al cuore dell'Unione europea e della sua moneta. Basta ricordare ciò che hanno fatto il presidente Prodi e il presidente Napolitano e tanti altri. Ricordo quanto il Partito Democratico abbia portato responsabilmente l'onere politico, così come del resto Forza Italia, in un momento molto difficile per il Paese che ho vissuto da vicino. Non possiamo fare a meno di creare dei piccoli strappi che - poi - vengono moltiplicati nelle cronache interne e, soprattutto, nei riporti che vengono fatti all'estero? Perché gettare sassi nello stagno che non hanno seguito, ma che turbano? Non si vuole il *fiscal compact*? Si vuole tornare al Trattato di Maastricht? Si dica esattamente che cosa si intende, lo si discuta con i potenziali alleati, ma non si lasci il mondo e i mercati nella sensazione che l'Italia non abbia ancora veramente assimilato la cultura di una certa disciplina di bilancio, che pure ha sottoscritto. Ieri non sono stato tanto sorpreso del fatto che il Capogruppo del Partito Democratico abbia promosso una mozione sul tema importante e delicato della Banca d'Italia. Sono stato, viceversa, molto sorpreso del fatto che 213 deputati si siano sentiti di approvare quella mozione. Ci rendiamo conto, senza entrare nel merito delle persone, che sono temi che tra l'altro riguardano inestricabilmente anche l'Europa, perché la nostra Banca d'Italia fa parte del sistema europeo delle banche centrali? rendere la testimonianza - qualunque cosa uno pensi sul complicatissimo tema bancario - del fatto che il Governatore della Banca d'Italia, e il 2012 (era l'attuale Governatore della Banca d'Italia, con i suoi uomini), ha avuto un ruolo fondamentale, di concerto con il Governo e senza minimamente intaccare l'autonomia della Banca d'Italia nel sistema europeo, per portare per portare sui tavoli europei la proposta dello scudo anti-*spread*, senza la quale non ci sarebbe stata neppure la successiva evoluzione, molto aperturista, della Banca centrale europea, dalla quale l'Italia ha preso la benedizione di una manna che forse erroneamente pensiamo destinata a non terminare mai. Il ruolo della Banca d'Italia in questo è stato molto importante. Concludo dicendo ci sarà presto l'occasione per avere vivacissimi dibattiti sul tema europeo: mi riferisco alle elezioni europee del maggio 2019, che il presidente Gentiloni Silveri ha richiamato. Non possiamo, da qui ad allora, cercare di corrispondere al suo auspicio di presentarci di presentarci più uniti e senza controversie, che comunque sono fuori tempo e che non potrebbero avere effetto concreto, per lasciare, noi come Italia, una maggiore traccia in Europa? e di ciò vorrei rallegrarmi con il Presidente e con i suoi collaboratori. Mi trovavo la settimana scorsa a Sofia, in un incontro con il Primo Ministro bulgaro, che - com'è noto - assumerà dal 1° gennaio la funzione di Presidente ruotante del Consiglio Non ho perso l'occasione per fare un riferimento a EMA, ovviamente, e ho visto come anche in quel punto della periferia d'Europa la preparazione fosse molto approfondita. Non tocca a me dire se ci siano state o meno conversazioni e accordi tra i due Presidenti del Consiglio. Con quella stessa unità, interpretando anche l'auspicio del Presidente, io credo che sia interesse di noi tutti fare questi quindici mesi, anche se ci sono di mezzo le elezioni italiane, in apnea rispetto a dibattiti viscerali europei. del Consiglio, cercherò di essere sintetico, perché è un'abitudine importante quella che lei venga a riferire a noi prima del Consiglio europeo ed è importante che noi corrispondiamo alla stessa abitudine esprimendo le opinioni dei nostri Gruppi senza indugiare molto. Anzitutto io confesso una certa preoccupazione. Il presidente Monti la proiettava, in particolare, per le nostre domestiche vicende, su cose che che certamente sono destinate ad acuirsi durante la prossima campagna elettorale, per cui capisco questo aspetto. Io aggiungo la preoccupazione per uno scenario europeo che temo, a fronte delle grandi questioni che l'Europa deve oggi risolvere, difficilmente potrà corrispondere con un equilibrio politico in grado di farle fare dei passi avanti. Spero di sbagliare naturalmente. Temo che il nuovo Governo tedesco finirà per essere maggiormente in difficoltà rispetto alle grandi scelte che dalla Germania l'Europa si attende e temo che le tante elezioni politiche locali, così come si è visto in Austria, facciano emergere quello che difficilmente può ricevere degli applausi italiani. Gentiloni Silveri si meravigliava; si meravigliava; anche io mi meraviglio di tanti applausi senza freni, magari sul nominalismo dell'appartenenza ad un partito popolare europeo che purtroppo - lo dico io che sono un popolare europeo da sempre e lo sarò per

finiscano inevitabilmente per creare dei problemi al mio Paese, l'Italia, che è impegnata più di qualsiasi altro Paese nel fronteggiare una

ha fatto accordi per cercare di rafforzare il dispositivo di guardia frontiera libica; il Ministro dell'interno ha fatto accordi con le municipalità libiche. Il risultato di tutto questo è un calo vertiginoso delle migrazioni,

come rappresentativo di un'Italia che non è stata a guardare, ma nell'indifferenza europea. Diciamoci la verità: mentre l'Europa, grazie alla spinta della Germania, è riuscita a realizzare un accordo economico forte con la Turchia, noi non abbiamo avuto la stessa capacità, ma abbiamo dovuto fare da soli. Oggi giustamente il Presidente del Consiglio chiede chiede il mandato a questo Parlamento per andare in Europa, al Consiglio europeo, chiedendo ai *partner* un aiuto sulla politica mediterranea. Questo aiuto non è dato all'Italia, checché se ne possa pensare, ma all'Europa stessa; infatti, o noi riusciamo a risolvere questo problema di concerto con i nostri *partner* europei, oppure inevitabilmente anche loro finiranno per avere ripercussioni negative. occorre prioritariamente un rafforzamento della politica mediterranea. L'Europa per troppo tempo ha guardato, anche giustamente, a Nord‑Est e oggi deve stabilire che c'è una priorità:

si sta prefigurando un *hub* del gas importante, con collaborazioni inedite tra Paesi come Cipro, Israele, Egitto, Paesi di segno, tradizioni, storie diversi. C'è tanto da fare e l'Europa deve assecondare il *focus* sul Mediterraneo. Secondo punto: la *web tax*. Sono totalmente d'accordo. Tutti noi vediamo le nuove tecnologie del *web* come grandi opportunità per i nostri Paesi; tutti noi riteniamo che la globalizzazione, anche da questo punto di vista, abbia portato a noi delle possibilità che in passato non c'erano. Ma noi dobbiamo evitare che i governi siano succubi dei giganti del *web* dare loro la possibilità di fare semplicemente a livello europeo quello che è giusto che facciano, cioè tassare questi grandi giganti, che oggi sono molto più potenti di molti Stati del mondo e dettano le regole. Non in Europa.

ma se l'Europa non recupera, sul piano della politica estera e della difesa, una dimensione comunitaria più forte, ogni sforzo di integrazione fallirà.

che le Nazioni Unite avevano insediato, c'erano altri attori principali della politica europea che lavoravano per la tripartizione della Libia. Oggi, sul tema della politica di difesa

non ci possono essere equivoci. Il Regno Unito è una ricchezza per l'Europa, rimarrà europeo anche fuori dall'Unione europea è bene che rivendichiamo parità di trattamento anche per i nostri connazionali che si trovano in quel Paese. Io penso che, con buona volontà, ci si possa intendere con gli amici della Gran Bretagna, perché anche loro oggi, sospinti dal vento del populismo, che prima fa nascere messianiche attese e poi sempre questo bisognerebbe pensare anche per il futuro in Italia)*,* si trovano a non saper più che direzione di marcia prendere. pertanto questo nostro atteggiamento di amicizia e cerchiamo di essere *partner* attivi in un negoziato che deve prendere il volo, perché è necessario chiarire la dimensione del rapporto e della *partnership* tra Unione europea e Regno Unito.

i prossimi anni saranno quelli decisivi per l'Europa, un'Europa che non sappiamo come sopravvivrà, che forse si allontanerà dai valori

questo è un passaggio ed un momento decisivo. La paura, o quanto meno il timore che noi abbiamo è che l'Italia e il suo Governo non siano in grado di dettare l'agenda che ci interessa;

Theresa May parla di 20 miliardi, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani parla di 50-60 miliardi, il «Financial Times» parla di 100 miliardi.

una trattativa in base alla quale il Paese che esce abbia più vantaggi dei Paesi che rimangano. Noi siamo qui a ottemperare alle regole imposte dall'Europa e addirittura trattiamo al ribasso - perché di questa cifra non si è parlato - l'uscita della Gran Bretagna.

dell'austerità, coniugata con la flessibilità. Siamo tanto lontani che, addirittura, un funzionario, tale signora Danièle Nouy, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE, stabilisce nuove regole per le banche italiane.

si è sentito in dovere di ricordare che la BCE non è una monade che agisce in un vuoto pneumatico e ha invitato la signora Nouy a tenere conto del fatto che il legislatore in Europa sia un altro. Mi auguro, quindi, che anche di questo parlerete nei prossimi giorni in Europa. però, sulla Libia che vorrei focalizzare la maggiore parte del mio intervento. C'è stato disinteresse dell'Unione europea. L'Europa si è girata dall'altra parte, salvo quando si è trattata della Turchia: tre miliardi sono subito arrivati

Bene, non solo è accaduto che l'Europa e i Paesi europei si siano girati dall'altra parte, ma è anche avvenuto che alcuni Paesi - lei sa bene a cosa mi possa riferire - sono intervenuti contro gli interessi italiani.

scritto e il suo Governo ha accettato che l'Esecutivo si impegnava a operare a livello diplomatico nelle opportune sedi internazionali e nell'ambito delle relazioni bilaterali affinché nessuna iniziativa unilaterale non coordinata potesse pregiudicare l'efficacia della missione. Detto in parole molto povere, si voleva dire: noi dobbiamo far fronte a un problema che ci riguarda direttamente; sappiamo che l'Europa si é girata dall'altra parte e chiediamo all'Europa che nessuno intervenga. Invece è accaduto. A Sabrata - lei forse lo saprà - il Governo legittimamente, oltre a parlare con il Governo Sarraj o con Haftar, che è stato ricevuto, parla anche con le milizie sul posto. Le milizie, che ci hanno anch'esse aiutato, oltre alle altre iniziative, a interrompere o ad attenuare il flusso della migrazione economica dalle coste libiche, oggi sono state battute sul campo da altre milizie che, guarda caso, sono supportate da Servizi di altri Paesi europei. Ciò vuol dire che in quella sede questi temi vanno posti; non è possibile immaginare che si compia uno sforzo colossale, in termini di miliardi per i contribuenti italiani e in termini di accordo complessivo per il sistema italiano rispetto a questo fenomeno e poi i Paesi alleati si permettano sul campo di contrastare e contraddire

Allora, dobbiamo stare attenti che quegli stessi *foreign fighter*, che stanno scappando dalle aree che il Governo siriano, i curdi, i russi e gli iraniani stanno cercando di occupare, anche a beneficio della nostra collettività e comunità, non arrivino sulle coste italiane. *(Applausi

che la Commissione difesa, su nostro stimolo e iniziativa, ha svolto un'indagine conoscitiva su ciò che facevano le ONG; che è stato dimostrato e certificato che quelle ONG a 12 miglia dalle coste libiche fossero un fattore d'attrazione (tecnicamente e che consentissero di incrementare il numero delle partenze, ma anche di morti. Lei non ha nemmeno ricordato quello che cercavo di accennarle prima, cioè che abbiamo contribuito largamente a che il suo Governo potesse disporre dell'autorizzazione a partire dalle coste, a bloccare le coste. In questo scorcio di legislatura abbastanza confuso (quello che è successo ieri in Aula alla Camera

soli*. Non so quanti di noi o di voi abitualmente guardino le statistiche e si chiedano chi sono coloro che sono arrivati sulle coste italiane.

c'è certezza, dovremmo affrontare adesso una discussione sullo *ius soli* a favore di 800.000 persone che frequentano un ambiente familiare nel quale non sappiamo quale sia il grado di amore, di affezione, di riconoscimento delle regole della nostra comunità. Signor Presidente del Consiglio, mi rivolgo a lei perché cita spesso questo argomento, verifichiamo la voglia che hanno quelle persone, che ha quell'ambiente familiare di riconoscersi nella nostra comunità, nella nostra storia, nelle nostre tradizioni, nelle nostre regole, nella voglia di appartenenza alla nostra comunità se questo non accadrà, come temo, sarà largamente prevalente il fatto di dare la cittadinanza a persone, bambini, minori, ma anche persone più grandi che non si sentono e non vogliono essere e sentirsi italiani.

Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio, colleghe e colleghi, malessere europeo è la definizione uscita dalla penna prestigiosa di Claudio Magris, un autore che ci ha narrato la civiltà letteraria della Mitteleuropa. Se Parigi, come si è detto, è stata la capitale del XIX secolo, Vienna è stata la capitale culturale del XX secolo. Lì l'Europa si specchia ancora e ancora rivela il suo volto e per questo, dopo la Germania, l'Austria ci dà un altro segnale inquietante. Leggo così, signor presidente Gentiloni Silveri, quello che lei chiama "momento di transizione", o "fase contraddittoria" dell'Unione europea. Proprio nel momento in cui i flussi migratori sembrano non presentarsi più come un dramma da stato d'eccezione, proprio ora la reazione popolare, soprattutto elettorale, si fa più virulenta. L'abbiamo visto nel Regno Unito, poi in Francia, adesso nel cuore dell'Europa. Ha ragione forse chi sostiene che meno il disagio sociale e più una sorta di disagio esistenziale è la vera causa scatenante. O forse è meglio dire che si scaricano lì, sulla paura del diverso e dell'estraneo, tutte le quotidiane difficoltà materiali delle persone. persone. Evidentemente il problema - l'immigrazione vista come pericolo - si è radicato nella coscienza, si potrebbe dire nel subcosciente, di una parte consistente di opinione pubblica. Questa falsa apparenza va smascherata: combattendo a viso aperto quelle forze politiche che su questo tema pensano di far fruttare il loro consenso. Però - e questo mi interessa più di dire dobbiamo sapere, e capire, che un sentimento di insicurezza, di incertezza, e addirittura di paura, esiste come dato di realtà, soprattutto nelle fasce di popolazione e negli spazi di territorio (penso alle periferie delle grandi città città metropolitane, ma anche ai piccoli borghi che si trovano a diretto contatto con la figura inedita e invadente a volte del migrante). Quel consenso che nasce dalla reazione contro quella figura va asciugato, con politiche mirate, con politiche intelligenti: innanzitutto - come lei ha molto sottolineato - a livello europeo. Occorre però che un gruppo, ristretto ma influente, di Paesi che più contano nell'agenda europea, prenda la testa di un'operazione di chiarimento a livello di massa su questo problema. E questo gruppo-guida non può che esprimersi in un asse italo-franco-tedesco: con misure pratiche concrete, ma anche e direi soprattutto, perché è quello che manca oggi, con una vera e propria offensiva culturale. Questi tre Paesi centrali, Italia, Francia, Germania, tutti e tre all'inizio di nuovi Parlamenti (come è all'inizio, in prospettiva, il nuovo Parlamento europeo) dovrebbero ognuno inaugurare una sorta di legislatura per l'Europa. L'Italia, come lei ha detto, per suo conto, non solo deve fare la sua parte ma la ha già fatta grazie anche alle iniziative del Capo del Governo in Europa e grazie alle politiche, appunto, di alcuni ministri,

si riesce a fare una buona politica. Questo è un insegnamento che dovremmo capire e far capire a tutti. *(Applausi in chiave europea, su quello che viene definito un epocale flusso migratorio, ma calcolando bene quantità e qualità dell'accoglienza, che vuol dire anche assicurazione di una sostenibilità finanziaria, finanziaria, civile, e di condizione umana, insieme a ragioni e tempi, i più rapidi possibili, del respingimento. Siamo confortati dalle recenti prese di posizione della Chiesa cattolica, che con il Papa e i suoi vescovi, sa in genere più di politica di tanti nostri nostri politici. Ma c'è un problema, colleghi e colleghe, forse meno pressante, ma ancora più importante, che non si può in questa sede approfondire ma vorrei che si trovasse il momento per farlo. Manca alle nostre istituzioni un luogo di riflessione e di confronto a livello, all'altezza, di cultura politica. Ed è tempo che si cominci a ragionare per la prossima legislatura su modi e tempi per costruirlo. Insomma, Insomma, siamo di fronte a questo paradosso: che un'Europa, nata e progettata per una vasta visione sovranazionale, si trovi oggi a fare i conti con spinte e pretese separatiste all'interno delle stesse Nazioni, con un moltiplicarsi di piccole patrie, con un micronazionalismo che sostituisce quello storico delle grandi Nazioni. Ora, qui bisogna fare attenzione: l'idea di Nazione affonda le sue radici nella storia lunga, appunto storia moderna. E stiamo vedendo quanto ancora essa sia capace di scaldare il cuore dei popoli; non a caso, dalla Serbia alla Catalogna se ne rivendicano le origini in antiche battaglie e in antiche date. L'idea di Nazione è un'idea storico-politica; come si può pensare di superarla proponendo un'Unione europea puramente economica, una sovranazionalità solamente monetaria, una globalizzazione solo di prodotti e non anche di produttori, cioè di lavoratori? anche le grandi, nazionalità, come unica passione di appartenenza rimasta a qualcosa per cui valga la pena. Sono rimasto impressionato dall'entusiasmo, dal calore, dai pianti di commozione delle folle catalane al pronunciamento della parola indipendenza. Alla secessione dalla propria Nazione si risponde con un progetto di oltrepassamento della Nazione stessa. Questo vuol dire più Europa. Per rovesciare questo neosovranismo, bisognerebbe tornare a pensare, e a ripensare, l'idea di sovranità, grande categoria della politica moderna, nei suoi sviluppi teorici, nei suoi mutamenti storici e nelle sue combinazioni future. Sovranità dei popoli è anche libertà, che va oltre l'individuo e attiene a una comunità, sempre più vasta e sempre più complessa. Signor Presidente, allora una vasta, ragionata, appassionata, operazione di educazione politica all'idea di Europa, simile a quella che avvenne sull'idea di Nazione. Bisogna ripartire dalle nuove generazioni, che sono già, direi per istinto, europee: non solo, come si dice spesso, tra quelli che circolano nel continente per via Erasmus, ma tra quelli, tanto più numerosi, che lavorano ormai nei Paesi europei, con mansioni spesso umili, o con attività a volte molto qualificate. Ma è necessaria un'educazione, una pedagogia a un sentire europeo. Uscirà nelle prossime settimane una raccolta di scritti e discorsi di Thomas Mann, dal titolo «Moniti all'Europa», tra l'altro con una intensa prefazione del presidente Napolitano. Moniti che salgono e ci raggiungono dal tragico Novecento.

Non è un autore di parte, è una delle più alte voci letterarie novecentesche. Le giovani generazioni non vanno retoricamente evocate come una risorsa già pronta per sostituire al meglio le vecchie generazioni. I giovani vanno

si deve pensare che ciò si può fare soltanto attraverso un'Europa politica. E l'Europa politica è un destino che ci attende; non dobbiamo aspettarlo, questo destino, dobbiamo progettarlo. E forse solo un grande balzo potrebbe essere la soluzione per superare questi piccoli passi che ci fanno stare praticamente fermi.

il Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre avrà luogo all'indomani delle elezioni politiche in Germania e in Austria. In ordine agli scenari futuri sono un po' più ottimista del presidente Casini, a proposito di tali elezioni,

(ÖVP), il Partito popolare austriaco, verso i Paesi di Visegrad o, ancora, verso destra, ma lavorerà nella migliore tradizione del Partito popolare europeo, per contenere il rafforzamento della destra europea. Ciò che è di fronte ai Paesi europei è l'esigenza di un nuovo patto europeo, in grado di proporre un sistema di governo dell'euro, nel quale responsabilità e condivisione dei rischi siano punti irrinunciabili, in una visione economica che non sia segnata da ulteriori vincoli restrittivi per i Paesi che dimostrino una reale capacità di stabilizzazione dei conti pubblici, come l'Italia. Diversamente operando, si metterebbe certamente a rischio la ancora fragile e non consolidata ripresa economica in tanti Stati membri. Restiamo anche convinti che l'unica risposta al populismo sia un'Europa più forte, che dia spazio a Regioni e comunità autonome, con un rafforzamento delle istituzioni europee, per avviare una politica di difesa comune e, sul piano economico, per istituire un Ministro delle finanze europeo, con il rafforzamento anche del ruolo della Banca

di dimostrare solidarietà e di rispettare le sentenze della Corte di giustizia si comportano in modo assolutamente inaccettabile, negando ogni principio di solidarietà. Condividiamo anche la valutazione del Presidente del Consiglio in ordine alla Brexit. Le proposte del Governo britannico per rispettare i propri obblighi finanziari e i principi e gli obiettivi di protezione dei

del fondo europeo, la riforma del sistema di asilo e l'attuazione del sistema di riallocazione dei profughi. Per attribuire un accettabile livello di credibilità a tale dibattito è necessario

Condividiamo inoltre l'impegno del Governo Gentiloni Silveri affinché il confronto sulle imprese digitali e la *web tax* sia ispirato al principio che la tassazione dei profitti avvenga dove essi sono stati creati. Mi permetto però di segnalare al Presidente del Consiglio e, in questo caso, al sottosegretario Gozi un altro tema che purtroppo il Presidente del Consiglio non ha affrontato nella sua relazione e nelle sue comunicazioni, che per il resto abbiamo molto Pensiamo infatti che le istituzioni europee non dovrebbero mantenere l'attuale posizione, molto defilata, sulla questione catalana, nascondendosi dietro lo stereotipo che si tratti di una questione interna allo Stato spagnolo. Pensiamo invece che in una comunità, come è l'Europa, le crisi istituzionali interne di ciascuno Stato membro interessino tutti i membri della comunità. Se in una famiglia, come è quella europea, un componente non riesce a risolvere un problema, è naturale che i familiari si interessino e non si voltino dall'altra parte, fingendo di non vedere, attualmente facendo, purtroppo, le istituzioni europee e anche gli altri Stati membri. Nel caso della Catalogna, infatti è di tutta evidenza l'inadeguatezza dell'attuale Governo spagnolo, in particolare del presidente Rajoy. È stato Rajoy e il suo Partito Popolare a essere il principale responsabile dell'accentuazione di questa crisi. Ricordo infatti che sono stati loro a far saltare l'accordo, faticosamente raggiunto nel 2005, tra il Governo del presidente Zapatero e le autorità catalane. È stato il Partito Popolare a presentare il famigerato ricorso alla Corte costituzionale, che poi ha portato alla cancellazione delle modifiche dello statuto della Catalogna. Questo ricorso si è però rivelato un'autentica vittoria di Pirro: pensavano di essere astuti, ma hanno causato la più grande crisi dello Stato spagnolo nel periodo *post*-franchista, spingendo per molti anni, con la negazione di ogni dialogo, anche le forze moderate spagnole verso il separatismo, benché la stragrande maggioranza dei catalani non voglia la secessione, ma un'autonomia più forte.

evidentemente siamo particolarmente sensibili a questo tema, anche perché è facilmente immaginabile cosa sarebbe successo a noi in Alto Adige-Südtirol, qualora la Corte costituzionale

non avevamo un Mariano Rajoy, ma c'erano personaggi lungimiranti come Aldo Moro, Giulio Andreotti, Alcide Berloffa e Silvius Magnago, per citarne solo alcuni, e l'Italia ha dato un ottimo esempio di come si affrontano efficacemente le crisi interne: non gettando continuamente benzina sul fuoco, ma con la strada del dialogo. Solo così è stato possibile superare un passato doloroso e dare concreta risposta alle legittime richieste delle popolazioni locali di maggiore autonomia. La soluzione non è quindi la prova di forza, la politica del manganello e la repressione antidemocratica alla Rajoy e nemmeno la secessione, ma la trattativa e il negoziato. L'Italia,

il Governo spagnolo avvii una costruttiva trattativa politica con i rappresentanti della Catalogna allo scopo di concedere forme più ampie di autogoverno, come del resto la stessa Spagna ha già concesso ai Paesi baschi.

Presidente, qui ci riempiamo la bocca di Europa, di Unione europea, di Consiglio europeo, con la legge elettorale liberticida, che state liquidando come affare di bottega tra soci in affari, spingete l'Italia su una deriva antidemocratica che ci porta fuori dall'Europa civile. fantasma e contumace, potrebbe essere l'ultimo Presidente del Consiglio a sedere al Consiglio europeo. Le sembra una provocazione eccessiva? Immaginate che Francia, Spagna, Germania o Regno Unito cambino le loro leggi elettorali a sei mesi dalla scadenza della legislatura, solo e soltanto per danneggiare una forza politica. Vi immaginate le reazioni? Bisogna ricordare che il codice di buona condotta in materia elettorale del Consiglio d'Europa del 2003, all'articolo 65: recita «ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno)». Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito». Anche in relazione a questo documento, la Bulgaria venne censurata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per aver modificato la legge elettorale in queste condizioni. La Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 348 del 2007, ha assunto le norme CEDU (e dunque il Codice di buona condotta summenzionato) come «fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all'articolo 117 della Costituzione». la volontà di manipolare è manifesta nelle candide ammissioni del condannato Berlusconi, ma anche nelle parole e opere del Presidente del Consiglio. Nel suo discorso programmatico, nel dicembre 2016, lei ebbe a dichiarare che il Governo avrebbe cercato di accompagnare, di facilitare il confronto sulla legge elettorale, senza esserne l'attore principale. Il Governo ha fatto peggio, infatti: si è nominato regista di un film dell'orrore e pure interprete nel ruolo dell'assassino; assassino del confronto e del dibattito ponendo alla Camera tre fiducie illegittime (e altre sono annunciate qui). Sono illegittime perché non rientranti nel programma di Governo, come da lui stesso dichiarato.

io toccherò un solo punto. A me va bene che il Presidente del Consiglio sia partito, perché il sottosegretario Gozi conosce benissimo il lavoro che abbiamo svolto con il Comitato per le questioni italiani all'estero. Io parlo nella veste di Presidente di tale Comitato, una veste da sempre stropicciata, come sa il ministro Finocchiaro, direi in questi giorni stracciata dalla legge elettorale; però porto sempre questa veste. Il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha svolto una rapida indagine per tentare di capire gli effetti che la Brexit rischia di provocare sui nostri concittadini che vivono in Inghilterra. Vorrei ricordare che circa 600.000 italiani sono oggi residenti in Inghilterra, ma questo tema riguarda 4,5 milioni di cittadini europei,

che riassumo con un solo concetto. Ho apprezzato che il Presidente del Consiglio abbia detto che devono essere difesi tutti i diritti dei nostri cittadini. Siamo perfettamente d'accordo con questo ma, in realtà, noi chiediamo al Governo italiano di portare in Europa una riflessione sulla strategia di fondo che l'Europa sempre ha avuto nei negoziati con Paesi terzi. L'Europa ha sempre avuto come linea: negli accordi si prende tutto o non c'è niente negli accordi. Porto l'esempio dei dodici accordi tra l'Unione europea e la Svizzera: il tutto o niente è stata una linea giusta, perché ha obbligato la Svizzera ad accettare l'accordo sulla libera circolazione delle persone, quando loro erano interessati agli accordi finanziari e sulle merci. Dunque il tutto o niente in un negoziato con un Paese terzo va benissimo. noi non possiamo accettarlo; qui noi dobbiamo assolutamente avere l'impegno che il tema dello *status* dei nostri milioni e mezzo di cittadini europei sia definito al più presto. Uso una parola che non è mia, una parola brutta: «ostaggio». Questa parola è stata usata da Michel Barnier quando è venuto qui in Senato e questa parola l'abbiamo sentita più volte negli incontri con le nostre comunità in Inghilterra. Noi non possiamo accettare che si vada a questo negoziato con la tecnica classica del tutto o niente. Qui deve essere definita la situazione dei nostri cittadini nel rispetto

su questo non c'è dubbio e io condivido pienamente l'intervento del Presidente del Consiglio. Però, non ci basta la risposta che il tema dei cittadini è una priorità: deve essere assolutamente trattato prima di tutti gli altri temi e concluso alla data di scadenza naturale dei negoziati, in quanto nessuno oggi è in grado di dire in che modo arriveremo a quella data con l'insieme del negoziato.

Possiamo demonizzarla e dire che tutti i problemi del mondo provengono dall'Europa. Qualcuno, però, ci ha detto: «L'Europa è come l'aria; ci accorgiamo che è vitale quando ne sentiamo la mancanza».

ha tratteggiato la difficoltà di questo negoziato sulla Brexit, un po' nei termini che venivano anche evocati prima di me dal collega Micheloni e che, in qualche modo, ha portato all'attenzione della Commissione affari esteri, emigrazione del Senato il negoziatore dell'Europa Barnier. Francamente, rispetto a questo minuetto sui quattrini ma avendo l'eleganza di differire il momento in cui si tratterà davvero di quattrini - a me, che non sono mai stato un suo ammiratore, veniva in mente, con qualche nostalgia,

prendendo per la giacca Emilio Colombo e Gianni De Michelis al grido di: «*I want my money back!*». Quella brutalità, rispetto a quell'ipocrisia da minuetto viennese, non è un motivo per guardare, neppur "tutto sommato" con soddisfazione, questa stagione di transizione europea: tutto è confuso e nulla va nella direzione di una maggior forza dell'Unione europea.

si è rivelata un disastro e non per pettegolezzi sull'alto tasso etilico del presidente Juncker, cui ha fatto bene il Presidente del Consiglio a esprimere gratitudine per le espressioni adoperate nei confronti del nostro Paese. Ma a che titolo Juncker dice al Parlamento europeo che, tanto, la Turchia è comunque fuori da ogni possibilità di entrare in Europa? Se ha titolo a dirlo, lo ripetesse, per esempio, domani al Consiglio europeo, altrimenti non ha senso. E che dire della Vice Presidente, la tanto accondiscendente Mogherini? Nei giorni scorsi, in mezzo a tante contraddizioni, il presidente Trump, in modo meno scomposto del solito, ha detto al mondo qualche cosa di abbastanza chiaro,

era stato tutelato dalla Presidenza Obama per otto anni, almeno per l'America volge al termine. E la Mogherini non si è accorta di niente! Ieri a Teheran l'ho sentita fare l'elogio

hanno ammazzato 30.000 persone e usano la tortura e la pena di morte con libidine. Come facciamo a non cogliere come europei tali questioni? A settembre presso le Nazioni Unite, qualche esponente sovranista, ma la Fondazione Danielle Mitterrand, a nome del Comitato diritti umani, ha citato sette di questi gentiluomini iraniani come gotha della criminalità. Perché la Mogherini è all'inseguimento di un ruolo pseudodiplomatico, o comunque televisivo, al seguito di una priorità della politica americana che non c'è più? Da questo punto di vista, la Commissione europea è veramente qualcosa di opaco, di insistente, di deludente, che vive in un mondo tutto suo. Mi si consenta un'ultima considerazione. Mi auguro che domani il Presidente del Consiglio italiano riesca a farsi valere e a convincere su tutti gli argomenti che ci ha detto; ma questa Europa a 28 - che diventano 27

e non affrontiamo invece il tema che la politica dell'allargamento, una politica voluta dall'allora presidente dell'Unione Romano Prodi, è stata talmente scombinata

il Governo italiano non smentisce il capo della marina militare iraniana, che, insieme ai militari iraniani, ieri a Venezia parlava, in un simposio, di cooperazione iraniano‑italiana? Di queste "mogherinate" né l'Italia, né l'Europa hanno alcun bisogno. Signor Presidente, è con un certo imbarazzo e con una certa difficoltà che interveniamo durante questa discussione. Il primo motivo è legato al fatto che al fatto che il Presidente del Consiglio è apparso in questa seduta, ha fatto il suo intervento e poi se n'è andato, con una presenza del Governo che ormai è molto limitata, con un rito ormai stanco, quello delle comunicazioni del Presidente del Consiglio prima dei

una situazione molto semplice: o l'attuale Governo è totalmente fuori dalla realtà o state ancora tentando vanamente di prendere in giro gli italiani rispetto a quella che è la reale situazione del nostro Paese. Il Presidente del Consiglio ha parlato di successi dell'Italia, con un ottimismo e un atteggiamento che - come ho detto prima - è molto lontano da quella che è la vera situazione che stanno vivendo i cittadini tutti i giorni. Cercherò di portare semplicemente alcuni dati e alcuni numeri, per dimostrare che questo ottimismo e questo atteggiamento sbagliato da parte del Governo è evidente, è chiaro, è innegabile. innanzitutto al tema dell'immigrazione, che sarà uno dei temi che verranno trattati. L'anno scorso c'è stato un arrivo di migranti in Italia superiore a 170.000 unità. Ora ci troviamo nel mese di ottobre, ma i dati dicono che a fine settembre gli arrivi ammontavano a quasi 200.000 unità, con un *record* assoluto rispetto agli ingressi e quindi con una totale incapacità di questo Governo, sia in sede italiana italiana sia in sede europea, di arginare questo fenomeno. I numeri parlano chiaro e non possono essere controvertiti da atteggiamenti ottimistici da parte del Ministro dell'interno o del Presidente del Consiglio.

con un +15,4 per cento rispetto all'anno precedente. Quindi stiamo vivendo in una fase molto grave della storia di questo Paese, in cui siamo capaci di attrarre migranti da tutti i Paesi del mondo, senza arginare questo fenomeno, e stiamo rendendo inospitale il nostro Paese a coloro che dovrebbero essere i protagonisti del domani, cioè le future generazioni.

Le nostre nuove generazioni stanno cercando fortuna all'estero e sono cacciate da questo Paese. Credo che questo sia uno dei dati più significativi, che evidenzia il fallimento di questo Governo e del precedente, rappresentato dal presidente del Consiglio Matteo Renzi. Sono cifre incontrovertibili, che non possono passare inosservate. Ma c'è un altro dato significativo. Coloro che emigrano, che scappano da questo Paese ormai inospitale, non vengono più esclusivamente dalle Regioni del Sud: il primato spetta alla Lombardia, con 23.000 cittadini che l'anno scorso sono partiti dal nostro Paese in cerca di fortuna; la seconda Regione è rappresentata dal Veneto, con 11.600 cittadini emigrati, che si sommano a quelli degli anni precedenti. Sono dati che dovrebbero preoccupare chiunque sia al Governo, che non dovrebbe avere al centro della propria azione politica la volontà di varare un provvedimento chiamato *ius soli*, per dare la cittadinanza a coloro che nascono qui a prescindere dalla loro effettiva appartenenza a questa nostra comunità. Dovrebbe essere un'altra la priorità di questo Governo e dei futuri Governi, che sicuramente cambieranno rotta, cioè quella di dare un futuro ai nostri giovani, di permettere alle nostre famiglie di crescere e di poter Stiamo assistendo alla distruzione di un modello culturale, quello europeo, che non è ostacolata da questo Governo, né dai Governi europei, ma è quasi incentivata. L'attuale Governo è complice di questi fenomeni. C'è un altro dato significativo che vogliamo mettere in evidenza: un sondaggio recente dimostra che solo il 36 per cento degli italiani considera un bene essere nell'Unione europea, a fronte di una media europea del 57

si è assistito al *referendum* della Scozia, che voleva staccarsi dalla Gran Bretagna, a quello della Brexit e a quello catalano, alle sconfitte elettorali dei partiti tradizionali europei, popolare e socialista, che sono ormai i guardiani del sistema e non rappresentano più i cittadini.

La richiesta di autonomia non è una contrapposizione tra regioni d'Europa o tra regioni d'Italia, tra popoli o tra comunità; è un'aspirazione all'autogoverno; è il segno di un contrasto tra i cittadini e lo Stato, tra i cittadini e i Governi centralisti. Governi che non sono più all'altezza di rappresentarli, che non li tutelano più, ma anzi li opprimono, ormai in modo insostenibile, con tassazioni, burocrazia, Signor Presidente, crediamo in un altro modello d'Europa, che non è quello che è stato portato avanti in questi ultimi anni dai Governi dal 2011 a oggi, e siamo sicuri che anche i cittadini italiani vogliano un cambiamento e lo esprimeranno in modo chiaro ed inequivocabile alle elezioni del prossimo anno.

Si tratterà quindi di questioni cruciali, insieme a quelle dell'immigrazione, della Brexit e delle altre richiamate dal Presidente del Consiglio, per il futuro dell'Europa. La strategia per il mercato unico digitale, adottata nel maggio 2015, deve essere infatti progressivamente ma rapidamente implementata con l'obiettivo di migliorare l'accesso ai beni e ai servizi digitali in tutta Europa per i cittadini e per le imprese e per cogliere a pieno il potenziale di crescita dell'economia digitale. Il Governo italiano ha già assunto un ruolo determinante, insieme ad alcuni *partner* europei, nella volontà di proseguire con decisione in direzione del mercato unico digitale. Contemporaneamente, il Governo italiano è impegnato ad accelerare e rafforzare la marcia per strutturare nel nostro Paese un adeguato ecosistema per l'innovazione digitale. Purtroppo siamo ancora, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi due-tre anni, in una situazione di svantaggio rispetto a molti Paesi dell'Unione. Il rapporto OCSE pubblicato pochi giorni fa colloca il nostro Paese in fondo alla classifica sul grado di avanzamento della trasformazione tecnologica. Non dobbiamo disconoscere questa realtà. Sono convinta che solo a partire dalla consapevolezza dei nostri ritardi possiamo meglio condividere la necessità di continuare un impegno per recuperare il tempo perduto. Il nostro Paese ha accumulato, a partire dall'inizio degli anni 2000, ritardi nella infrastrutturazione della banda larga, nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e del nostro apparato produttivo. Ciò ha determinato nel sistema pubblico una minore efficienza nella prestazione dei servizi a cittadini e imprese e nei settori della produzione una diminuita competitività ed una perdita di valore per la nostra economia. Un grave ritardo che abbiamo iniziato a recuperare negli ultimi tre anni, con una inversione di marcia davvero molto decisa, intrapresa prima dal Governo Renzi e poi dal Governo Gentiloni Mi riferisco, in particolare, agli investimenti ed alle misure previste dal piano per la banda ultralarga e dal piano Industria 4.0, che stanno dando una spinta straordinaria agli investimenti innovativi, alla digitalizzazione, agli investimenti in ricerca. In questi ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti: è cresciuta la consapevolezza dei benefici dell'innovazione e sono state adottate misure incisive per dare un adeguato supporto alle imprese, stimolando collaborazioni con università, enti di ricerca e *startup*. Non è necessario che mi dilunghi su questo punto, il Governo sa bene ciò che serve al Paese. Sono certa che condividiamo la convinzione che solo attraverso l'investimento nella scienza, nella tecnologia, nella ricerca e nell'innovazione possiamo dare slancio e rafforzare quella ripresa economica che significativi indicatori ci dicono in atto nel nostro Paese. La conferma, non scontata, nella manovra di bilancio per il 2018 della prosecuzione di Industria 4.0, che evolve in Impresa 4.0, il sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese, l'incentivo strutturale per l'occupazione giovanile, l'assunzione di 1.500 ricercatori dimostrano concretamente l'attenzione del Governo su questo fronte. L'innovazione digitale non è certo l'unico elemento, ma è sicuramente un fattore strategico per la crescita. Se però è vero che l'Italia è in ritardo nella sfida del digitale, è pur vero che complessivamente anche l'Unione europea lo è; in questo campo è ancora grande lo spazio di lavoro comune da affrontare. L'Europa è in ritardo, la politica tutta è in ritardo nell'affrontare le enormi questioni poste dalla rivoluzione digitale. Tuttavia, anche a livello europeo, nel 2016 e nel 2017 abbiamo compiuto passi in avanti davvero molto importanti. Mi riferisco alla questione della protezione dei dati, alla portabilità transfrontaliera dei contenuti *online* e, soprattutto, all'abolizione delle tariffe di *roaming* e all'accordo sull'accesso gratuito a Internet nei luoghi pubblici. Si tratta di misure molto concrete, che contribuiscono a migliorare la percezione di una Unione europea più vicina alle domande ed alle esigenze dei propri cittadini, in particolare dei giovani. Risposte utili anche a contrastare la falsa percezione, alimentata artatamente dalle forze populiste, di istituzioni e decisioni europee lontane dai problemi della vita reale degli europei. Per il futuro, la strategia dell'Unione si prefigge di espandere ulteriormente l'economia digitale. Secondo uno studio comunitario, il valore economico dei dati passerà in Europa dai 300 miliardi di euro del 2016 ai 739 miliardi di euro nel 2020. Le ultime Le ultime statistiche comunitarie ci informano inoltre di un aumento esponenziale degli attacchi informatici, aumentati del 300 per cento dal 2015, con l'80 per cento delle imprese europee che hanno subito almeno un incidente cibernetico nel corso dell'ultimo anno. Sono dati che mettono in evidenza, insieme all'urgenza di un quadro normativo adeguato, la necessità del completamento del mercato unico digitale entro il prossimo anno.

sistemi di istruzione e di formazione altamente qualificanti; maggiori investimenti in ricerca e sviluppo; un approccio comune in materia di sicurezza cibernetica e un aggiornato regime fiscale. Si tratta, insomma, di accompagnare e sostenere in Europa il processo in corso, nel settore pubblico così come in quello privato, perché nel mondo globale restare indietro nell'utilizzo delle nuove tecnologie connesse al digitale significa essere destinati alla irrilevanza. Nell'ambito degli enormi rivolgimenti dati dall'economia digitale emerge fra le questioni cruciali quella della sicurezza e della difesa, del controllo del fenomeno della radicalizzazione. Su questo piano i grandi operatori del *web*, che detengono a livello globale quantità enormi di dati, possono e devono collaborare con le istituzioni europee. L'attenzione dell'Unione europea rispetto alla sicurezza cibernetica è cresciuta molto, ma ora è il tempo di definire un quadro normativo uniforme.

Essa ha ovviamente ricadute economiche, ma anche un risvolto sul piano dell'equità: non è eticamente accettabile che ci siano imprese che non pagano le tasse, senza tralasciare le distorsioni sul piano della libera concorrenza e della competitività. si tratta di applicare anche all'economia digitale quel che vale per qualsiasi altro settore economico, il principio per cui le imprese devono pagare le tasse laddove producono i profitti. Voglio ricordare, a tal proposito, che gli enormi introiti che potrebbero derivare dalla *web tax* in Europa potrebbero essere utilizzati in modo proficuo per la formazione e la creazione di lavoro per i nostri giovani.

che è una base importante per l'integrazione europea. Non esiste futuro per il nostro Paese senza Unione europea, non può compiersi appieno l'Unione senza una sua piena realizzazione anche sociale e politica. Occorre più Europa, lo abbiamo visto bene, soffrendone le lacune, in occasione del grave dispiegarsi della vicenda catalana. A sessant'anni dalla firma del Trattato di Roma, di cui si è ricordato oggi l'anniversario, che istituì la Comunità economica europea, abbiamo il compito e la responsabilità

L'Europa che sta affrontando anche il tema della Brexit? Forse sarebbe il caso di levare la patente europea alla borsa di Londra perché è qui che si tratta il 70 per cento dei derivati sull'euro. Possiamo lasciare tutto questo nelle mani di uno Stato che non fa più parte dell'Unione europea? europea? Ultimamente persino il Fondo monetario internazionale ha detto che è opportuno un reddito universale per tutti, il reddito di cittadinanza che solo noi chiediamo. Ma allora di quale Europa stiamo parlando? Tra i tanti temi che si affronteranno nella nella riunione di domani, c'è anche quello della connettività. In Italia abbiamo alcune eccellenze che riguardano però solo alcune aree del Paese, tipicamente le grandi città. Questo lo afferma l'Agcom in un suo studio del 2017

Quindi, quando parliamo di questa infrastruttura in fibra parliamo di occasioni perse, volutamente perse, perché la realtà dei fatti è sempre la stessa. Negli ultimi vent'anni l'Italia su questo tema è ancora ostaggio degli accordi e dei compromessi al ribasso con l'imprenditore Silvio Berlusconi. Questo dovrebbe andare a raccontare al Consiglio europeo il Presidente del Consiglio, cioè che siamo vittime di un compromesso, di qualcuno che non ha voluto far sviluppare le telecomunicazioni in Italia.

tutti anche questo) il cui figlio è stato per lungo tempo responsabile economico del PD. Tutto questo sempre per continuare a difendere gli interessi economici di Berlusconi e quindi rinsaldare il patto d'acciaio tra il Partito Democratico e Forza Italia che ha bloccato questo Paese per vent'anni. Siamo ancora lì e anche la legge elettorale è frutto di questo accordo: è sempre questo che blocca lo sviluppo del nostro Paese sul tema delle telecomunicazioni. Se non ci fossero stati Berlusconi e le sue aziende a fare da stampella a questo Governo e a questa strana maggioranza, da tempo ve ne sareste andati tutti a casa.

il problema è sempre lo stesso perché è chiara la situazione in cui ci troviamo, è chiaro il fatto che il Presidente del Consiglio ormai è in scadenza e siamo tutti in attesa della legge elettorale, che tutti pensano porterà il Movimento 5 Stelle alla sconfitta. Eppure, come sempre, quando una legge è fatta contro qualcuno, quel qualcuno mostrerà la realtà di quei cittadini che sono veramente stanchi di questa consorteria che va avanti da venti anni.

sua e dell'Italia. Anche perché, signor Sottosegretario, l'Europa era composta da 28 Paesi, adesso da 27, ma non è coesa. Ci sono i Paesi baltici da una parte con i loro interessi e i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo che hanno tutt'altri interessi.

la prima fase non mi dilungo perché sull'Europa digitale, la difesa europea e la *web tax* avremo modo di discutere ma sul secondo punto, cioè sulle politiche migratorie comuni

capisce perché il suo popolo non lo comprende perché sui problemi dell'Europa si gioca una grossa partita. La nostra risoluzione è un

prendono tanto e altri, invece, non hanno nulla e sono in stato di povertà. Ecco che ne deriva che le condizioni essenziali per la concessione di aiuti e finanziamenti internazionali, il tanto vagheggiato "Piano Marshall", dovrà essere una forte spinta volta a favorire lo sviluppo democratico di quei Paesi. Signor Sottosegretario, è inutile che faccia riferimento al passato quando c'erano statisti che con quei Paesi dialogavano.

questo sacrificio, lo abbiamo fatto e ovviamente lo stiamo pagando noi. Non dimenticatevi Bettino Craxi quando dialogava con i palestinesi, non dimenticatevi Andreotti che riusciva a dialogare con l'Iran e con i Paesi mediorientali perché con quei Paesi bisogna dialogare, bisogna cercare di frenarli

sapere che l'Italia ha salvato l'onore dell'Europa e che siamo rispettosi dei diritti umani, ma bisogna anche dire che tutti questi immigrati che arrivano in Italia devono essere ricollocati non solo in Lombardia dove ne abbiamo la maggiore

con chi, invece, in maniera più accurata, ha voluto creare i presupposti per dare aiuti. Quindi noi riteniamo che nella nostra risoluzione ci siano gli spunti per far riuscire alla base a colmare il divario in termini di benessere complessivo. Abbiamo perciò inserito dei punti in cui il Governo deve rappresentare al Consiglio d'Europa l'entità degli sforzi fatti e prendere in considerazione considerazione l'attuale situazione economica e sociale dei Paesi di provenienza, che abbiamo ben illustrato nell'*incipit.* Il fenomeno deve richiedere altresì una maggiore partecipazione dei singoli Paesi europei nella ricollocazione dei migranti e nell'opera di rimpatrio dei non aventi nonché nel finanziamento degli oneri straordinari che derivano dal loro sostentamento e che non possono consistere nel solo riconoscimento di maggior margine di inflessibilità nel bilancio.

le parole pronunciate in quest'Assemblea erano e rimangono pietre e le pietre possono essere usate per costruire o colpire l'avversario. Il 14 dicembre 2016 il Presidente del Consiglio nel suo discorso di insediamento disse con chiarezza: «non vi è dubbio che quando quando discuterete - e il Governo darà il suo contribuito - le nuove regole elettorali, saremo tutti consapevoli che si tratterà di una discussione che inciderà sul modo di concepire il funzionamento della nostra democrazia. Questo credo sia un aspetto di cui certamente tener conto.

Ebbene non possiamo e non dobbiamo tacere su ciò che è accaduto in questi giorni e su quanto questi impegni siano stati traditi, divenendo carta straccia. Il Presidente del Consiglio si era impegnato di fronte al Parlamento, nell'atto del suo insediamento, a non invadere il terreno della legge elettorale che in tutto il mondo civile e avanzato è materia di competenza strettamente

Siamo di fronte - vorrei dirlo con forza, invitando tutti i colleghi di maggioranza e opposizione a riflettere - ad una chiara e grave alterazione della Costituzione materiale del nostro Paese. anzitutto ricordato che la nostra è una Repubblica parlamentare in cui il Parlamento sta sopra il Governo e non viceversa; è il Governo che riceve la fiducia dal Parlamento.

Un Governo che impone per la prima volta dal 1861, dall'Unità d'Italia, una doppia fiducia alla Camera e al Senato tradirebbe la Costituzione italiana. Questo Governo, che abbiamo lealmente sostenuto nei mesi passati in quest'Assemblea, non ha deluso solo noi, la nostra parte politica e il nostro Gruppo, ma tutti gli italiani che credono nella Costituzione italiana, nei suoi principi e nei valori espressi in quel testo.

Quale valore può avere il richiamo all'unità del Paese di fronte a fenomeni epocali, come quello dell'immigrazione? Un richiamo che viene da chi pochi mesi fa si era impegnato a tenere un comportamento costituzionalmente rispettoso delle prerogative del Parlamento

Colleghi! Senatore Fornaro, si rivolga alla Presidenza nel suo intervento.

Con questa sua scelta, il Governo ha indebolito anche la credibilità dell'Italia, perché in nessuna grande democrazia potrebbe capitare ciò che è capitato nel nostro Paese, parlamentari posti sotto il doppio ricatto della fiducia e della mancata ricandidatura da parte del loro capopartito, il tutto a poche settimane dalla fine naturale della legislatura. È in questa cornice di macerie nei rapporti parlamentari - prodotte dal Governo con tale scelta - che si svolge il dibattito sul prossimo Consiglio europeo.

ai temi dell'immigrazione, in breve, gli aiuti alla cooperazione internazionale vanno inseriti in progetti organici di sviluppo, coordinando meglio gli interventi dell'imprenditoria nazionale. Non possiamo però continuare a far finta di niente e a non vedere le violazioni dei diritti umani perpetrate L'Europa non deve continuare ad ignorare, nei fatti, il carattere strutturale delle migrazioni in atto senza una consapevolezza e una visione di lungo periodo si finisce solo per mettere la polvere sotto il tappeto, senza peraltro neppure rassicurare l'opinione pubblica degli Stati nazionali, come dimostrano le ultime elezioni in Austria. Infine, la tassazione

Ci vuole "il fisico" per competere con i giganti dell'economia digitale e affrontare gli impatti su diritti e occupazione dei lavoratori prodotti dalla cosiddetta un terreno nel quale l'Unione europea deve dimostrare di essere uno strumento utile ai cittadini e non uno strumento prono prono ai voleri delle *lobby* e delle multinazionali. Concludo, quindi, ribadendo la nostra profonda delusione nei confronti del Governo e delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, dopo la sua decisione di porre la fiducia

comunque per la sua relazione, che abbiamo ascoltato con vivo interesse, anche perché il Consiglio europeo, che si terrà il 19 e 20 ottobre prossimi, vede all'ordine del giorno alcuni temi, che ormai sono divenuti ricorrenti in questa Assemblea, ma che, a distanza dì quattro mesi circa dallo svolgimento dell'ultimo Consiglio europeo, a giugno, ha visto sensibili evoluzioni nelle situazioni politiche e iniziative di vari Governi europei, che sono certamente da valutare con la dovuta attenzione. Mi riferisco precisamente alla questione dei flussi migratori illegali e alle misure da adottare per controllarli. Signor Presidente, gli scenari delineatesi oggi in Europa non ci fanno star tranquilli, dal momento che in Germania la cancelliera Merkel ha vinto le elezioni politiche, ma il suo partito non è andato bene e ha perso tanti seggi in Parlamento, mentre il partito di estrema destra AfD ha sfondato, svolgendo una campagna di contestazione delle politiche sull'immigrazione e le scelte del Governo tedesco di accogliere migliaia di rifugiati provenienti dalla Siria e da altri Paesi a maggioranza musulmana. La Merkel, d'altro canto, che si prepara a fare i conti con un cambiamento della maggioranza, ha dichiarato apertamente che durante il nuovo mandato farà il necessario per capire le preoccupazioni, le ansie e le paure degli elettori che hanno scelto di votare AfD. Cosa questo significhi, credo che lo vedremo in un momento non tanto lontano. Nel frattempo, si è creata una coalizione di Stati in aperta opposizione ai migranti, formata da Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. In Austria abbiamo assistito alla recentissima vittoria di Sebastian Kurz, un Capo di Governo che sarebbe pronto ad allearsi con gli euroscettici del FPÖ, partito di Heinz-Christian Strache, il quale sembrerebbe tentato dall'idea di fare asse con la coalizione antimigranti e quindi di continuare ad ostacolare le politiche di accoglienze dell'Unione europea. Questi Paesi, infatti, cui aggiungo adesso anche la Germania, sembrano preoccupati dal problema della riconquista della fiducia dei propri cittadini che sembra passare proprio dall'abbandono delle politiche di accoglienza di Bruxelles e potrebbero essere tentati dall'idea di smarcarsi dai concetti di mutualità, sia in campo economico che migratorio. Se anche l'Austria dovesse apertamente appoggiare la coalizione antimigranti capeggiata dall'Ungheria, assisteremmo veramente a un proliferare del fenomeno della blindatura dei confini sia interni che esterni. Inoltre, non dimentichiamo che la settimana prossima andrà al voto la Repubblica Ceca, dove gli osservatori dicono di attendersi la vittoria del partito euroscettico ANO 2011, guidato da Andrej Babis. Quindi, possiamo dire che in Europa spira un vento sinistro, bieco, che rinfocola scetticismo e precarietà: un vento che alimenta le paure dei collegamenti tra immigrazione e terrorismo, che rifiuta le quote obbligatorie di accoglienza decise dall'Europa, poiché sostiene che questo è un sistema che incentiva i flussi migratori e corrobora pure gli affari dei trafficanti. Un vento che si trasforma quando raggiunge le piazze e le periferie del Continente in *mainstream*, favorendo la convinzione che le persone non possono essere trattenute in un luogo qualsiasi contro il loro volere. Soprattutto, è un vento che spinge sul concetto di sovranità, sostenendo che nessuno può comprimere il diritto di uno Stato nazionale di decidere cosa fare sul proprio territorio, allorché la volontà popolare e il senso comune si atteggiano in modo contrario alla volontà di Bruxelles. Dico questo, signor Presidente, perché mi sembra che il cambio di rotta che stiamo osservando depotenzi le politiche europee con il rischio che si creino manovre tali per cui l'Italia potrebbe trovarsi ancora più sola ad affrontare il fenomeno migratorio, di fronte alle spinte che anche qui da noi fanno appello alla sovranità e all'interesse nazionale. nazionale. Il Presidente del Consiglio ha detto che in tema di flussi migratori l'Italia ha salvato l'onore dell'Europa, ma lo ha fatto a spese dei cittadini italiani, dell'impegno delle Forze dell'ordine italiane, delle organizzazioni di protezione civile delle comunità locali italiane e delle risorse materiali Oggi abbiamo un'Europa che ha conosciuto il fenomeno Brexit, con la determinazione dell'Inghilterra di rendere più difficile persino l'afflusso di lavoratori europei. In Francia, Macron ha confermato di voler espellere i rifugiati che in Francia hanno commesso crimini. E poi c'è stata la vicenda della Catalogna, che pure si era distinta per le sue iniziative pro immigrati. è lo scenario che ci interroga oggi e su cui va fatta una seria riflessione. Le preoccupazioni per un ritardo nell'attuazione del piano del Governo per ridurre il flusso migratorio sono sono crescenti, così come crescenti sono i dubbi sulla possibile marginalizzazione dell'Italia rispetto al quadro europeo che si delineerà nei prossimi mesi. L'atteggiamento morbido, il lassismo, il pietismo ci hanno condotto a questa deprecabile situazione; ci hanno spinto in fondo al burrone. Altresì crescenti sono le perplessità per un Governo la cui volontà è quella di rafforzare

Abbiamo maturato il convincimento che la politica dell'Europa sul tema delle migrazioni non è mai stata compatta, univoca, chiara, ma ha subito continui cambiamenti di rotta, così come abbiamo spesso sentito in quest'Aula le lagnanze per alcune proposte dell'Unione europea fortemente sbagliate e inadeguate al fine di gestire una crisi così imponente. Dobbiamo renderci conto che queste criticità rendono ancora più fragile l'Europa. L'ho già detto in quest'Aula, signor Presidente e lo ribadisco: noi non siamo euroscettici, ma insistiamo fortemente sulla necessità di tutelare gli interessi del nostro Paese in tutti i settori, con 1'obiettivo di ridiscutere i nostri impegni in seno all'Unione. Non siamo euroscettici, ma europeisti convinti, sebbene critichiamo decisamente le *leadership* europee di oggi. L'atteggiamento rinunciatario della Commissione europea di non voler comprendere i deleteri fenomeni nel quotidiano, sul territorio, nelle periferie del continente,

piccolo Paese candidato all'adesione all'Unione europea, per incontrare i rappresentanti del Parlamento. Posso garantire che il quadro confuso dell'Unione europea desta non poche perplessità e indecisioni nei Governi dei Balcani, pregiudicando le politiche di allargamento. Insomma, signor Presidente del Consiglio, si impone un cambio di marcia serio e ci auguriamo che anche il Consiglio europeo nei prossimi due giorni ne senta la necessità; tuttavia, mi permetta di nutrire qualche dubbio al riguardo. Sicché, nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del del Gruppo cui sono iscritto, il Gruppo GAL, mi permetto di mostrare numerose perplessità sulle odierne comunicazioni.

e documenti di indirizzo, è del tutto ovvio che la discussione che oggi fa il Parlamento italiano abbia caratteristiche di pura ritualità: non c'è nessuna possibilità materiale e concreta per questo Parlamento di poter entrare non solo nelle decisioni del Consiglio europeo, ma nemmeno nel dibattito politico. A questo - come si può notare - va aggiunto il fatto che il Governo, forse anche per queste ragioni, si presenta a ranghi molto ridotti; è assente infatti il Presidente del Consiglio e questo fatto davvero la dice lunga su come il Parlamento venga tenuto in considerazione rispetto a scelte che invece meriterebbero ben altra attenzione e ben altra serietà. Devo dire anche, nel merito della relazione fatta dal presidente del Consiglio Gentiloni Silveri ( mi spiace che non sia qui), che francamente trovo un po' ingiustificato il suo ottimismo, se posso dire così, e lo dico, peraltro, anch'io da europeista convinto e da storico, per quanto riguarda me e il mio partito, fautore e sostenitore di posizioni europeiste. Credo, che se si fa finta di non guardare quello che è accaduto in Europa nel corso di questi anni e si fa finta di non guardare finanche quanto accade in queste settimane, davvero si rischia di commettere un errore politico con conseguenze molto molto serie. Si dice che abbiamo finalmente raggiunto un tasso di crescita stabile tra il 2 e il 2,2 per cento, dimenticando però di aggiungere che probabilmente questo risultato è dovuto a una congiuntura,

di una forte presenza e incremento di quelle forze politiche orientate verso la maggiore integrazione, proprio come se si facesse finta di non vedere quanto è accaduto politicamente, Sottosegretario, in questi anni nell'Unione europea. Come fate a non vedere che, invece, si sono affermate e continuano ad affermarsi, purtroppo, istanze molto diverse da quelle di cui parlate voi? Come fate, soprattutto, a non vedere che siamo dinanzi a un crollo politico delle forze politiche tradizionali, le forze *mainstream*, quelle che in tutti questi anni hanno fatto del *mantra* dell'Europa una sorta di paradigma indiscutibile? In questi anni in Europa è successo esattamente il contrario di quanto è stato raccontato: le forze politiche tradizionali sono quelle che, anche da un punto di vista elettorale, vivono maggiori elementi di difficoltà, mentre coalizioni di tutt'altro genere, che hanno maggiormente interpretato gli istinti di critica all'Unione europea, sono quelle che elettoralmente hanno ricevuto più voti. Ciò non è accaduto, fortunatamente, soltanto

come nella Spagna di Podemos, nella Francia di Mélenchon, nell'Inghilterra di Corbyn, nel Portogallo del Blocco di sinistra, dove, evidentemente, soggetti politici e sociali hanno in qualche modo detto che il re è nudo: Europa, l'ipotesi d'Europa che i principali Paesi europei hanno costruito in questi anni, che è stata un fattore generativo di gigantesche diseguaglianze sociali. A me veramente stupisce che in una

accenno a quello che oggi mina, con grandi elementi di contraddizione, le fondamenta di una possibile democrazia europea. Stupisce che non vi sia un accenno minimo al tema grande della democrazia, del *deficit* democratico, della mancanza della sovranità europea. Mi pare di poter dire che su questo davvero servirebbe una discussione molto più avanzata di quella che facciamo noi. Ancora, credo che questo ottimismo ingiustificato e questa rimozione di quanto accade intorno a noi i conti con l'altro grande elemento che invece andrebbe, una volta per tutte, messo al centro della discussione politica di questo Continente. O si prende atto fino in fondo che l'Europa così come è stata costruita, il vincolo dei Trattati, l'idea che l'unione monetaria dovesse venire prima di qualunque altro aspetto sono un fenomeno degenerato e degenerativo che provocherà inevitabilmente disgregazione e che non è semplicemente necessario, ma imprescindibile costruire elementi di radicale discontinuità rispetto a quanto è stato fatto nel corso di questi anni, oppure si assisterà in maniera supina e impotente a quella che, inevitabilmente, sarà una disgregazione. Noi ve lo diciamo oggi perché troppe volte, nel corso degli ultimi anni, abbiamo

nell'ordinamento europeo, divenendo giuridicamente superiore alla legislazione nazionale e rendendo in questo modo irreversibili le politiche di austerità. Capite o non capite che anche semplicemente un fatto come questo rischia di far diventare i dibattiti come quello che stiamo facendo stasera del tutto inutili rispetto a quello che potrà succedere nel corso degli anni che verranno?

Sottosegretario, che essa può introdurre degli elementi giganteschi di esautoramento della Commissione europea e, anche da questo punto di vista, di totale regressione rispetto a ciò che invece servirebbe? Mi pare che su queste questioni ci sia davvero da parte del Governo italiano e dei due principali Gruppi politici europei, quello socialista e quello popolare, uniti dallo stesso drammatico disastro elettorale che stanno compiendo in questi anni e dalla perdita di decine di milioni di voti di consenso, una gigantesca miopia nel non vedere quali sono i grandi elementi di fondo con cui bisognerebbe invece confrontarsi.

nel chiedere di conoscere fino in fondo la verità su quanto stabilito con questo benedetto Governo libico, su quello che sta accadendo sulla storia dei migranti su quello che accade sulle coste libiche (mi riferisco ai cosiddetti campi di concentramento presenti su quelle coste, dove vengono perpetrate torture e sevizie nei confronti dei migranti): su su questa cosa non si può consentire che possa esserci anche il minimo dubbio. Voi avete il dovere di dire fino in fondo cosa è stato stabilito dall'Italia, quali accordi sono stati presi, cosa è successo, se questi accordi riguardano soltanto la Libia, quali Governi sono stati tenuti

Domani, al Consiglio europeo, si parlerà anche di politica estera e di sicurezza comune, di progetto di difesa comune europea e anche di politica dell'immigrazione. Io ho preso appunti, signor Sottosegretario.

l'Italia spende circa 210 milioni di euro per queste sei missioni. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi su questa argomentazione, in modo tale che, se parliamo di difesa comune, prima partiamo dai presupposti di quello che è un modello di difesa italiano, dopodiché questo modello di difesa italiano lo portiamo a confronto con gli altri Paesi europei e potremmo magari tirar fuori da questo concetto di difesa comune qualcosa di conveniente anche per l'Italia. Ma così fino ad oggi non è stato. stato. Per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione, il presidente Gentiloni Silveri ha fornito una visione assolutamente fuori dalla realtà. Le riferisco un dato, relativo a questa mattina: questa mattina in Sicilia, a Trapani, è arrivata l'ennesima nave con circa 70 immigrati. È vero che il numero è sceso rispetto

Ebbene, occhio al lato destro del Mediterraneo (o sinistro, a seconda da dove lo guardiamo), cioè alla Tunisia, perché è quella la nuova via che si è aperta. Allora, questa visione ottimistica si scontra con la realtà dei fatti, che non può sicuramente sfuggirvi, perché sempre lo stesso Governo ha svenduto lo stesso Governo ha svenduto il territorio italiano per un pizzico di flessibilità e gli immigrati in quel caso sono arrivati giornalmente e a migliaia. Quindi ci sono decine di migliaia di immigrati che stanno sul suolo italiano

*(PD)*. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, ci sono quattro grandi questioni in agenda in questo Consiglio europeo, che sono anche le grandi sfide di questo tempo, in cui i temi dello sviluppo, della cooperazione, dell'innovazione e della sicurezza incrociano le opportunità e le difficoltà che abbiamo davanti a noi e che richiedono risposte sempre più veloci, efficaci e convincenti dell'opinione pubblica, su cui si misura anche la capacità della democrazia di essere una democrazia governante e non solo l'espressione di rituali parlamentaristici ormai desueti. Com'è già avvenuto tra le due guerre mondiali del secolo scorso, quando si interruppe la forte espansione del primo tempo della globalizzazione, assistiamo a ripiegamenti nazionalistici in politica e protezionistici nel commercio, vocazioni ingenuamente autarchiche in economia, vagheggianti improbabili orizzonti bucolici. Gli scambi commerciali crescono meno velocemente dell'economia per la seconda volta in centosessant'anni. La prima volta fu dopo la depressione del 1929 e l'ondata proibizionista che ne seguì. Il populismo e i nazionalismi non smettono di soffiare sull'Occidente, come il recente voto austriaco dimostra. In questo quadro l'Europa o si rafforza nella sua dimensione sovranazionale o rischia il suo dissolvimento, con tutto quello che ne consegue, soprattutto per i Paesi più fragili. Sulle questioni che questo Consiglio europeo dovrà affrontare (immigrazione, mercato digitale, difesa, relazioni esterne, Brexit) occorre quindi avere la piena consapevolezza della sfida che abbiamo di fronte. Non basta fare il punto su queste questioni. Sull'immigrazione è tempo di fare concreti passi avanti sulla riforma del sistema europeo comune di asilo e occorrono misure immediate aggiuntive, sia per controllare i flussi migratori illegali su tutte le rotte, sia per sostenere gli Stati membri in prima fila, come l'Italia, sia per rafforzare la cooperazione con le organizzazioni che operano sul campo, sia con il rafforzamento di Frontex. Ma non ci stancheremo di dire che occorre intensificare gli interventi di cooperazione verso il Nord Africa e l'Africa subsahariana che, senza una piena consapevolezza degli errori storici degli Stati nazionali (non dell'Unione europea) nei rapporti con l'Africa, che consenta di mettere in campo politiche di sviluppo e non di neocolonialismo, tali da risolvere il problema e non solo di contenerlo, noi non riusciremo a risolvere questi problemi epocali. Per fare questo occorrono, signori del Governo, signori del Parlamento, risorse aggiuntive nel bilancio europeo, senza le quali nessuno degli obiettivi enunciati può davvero essere perseguito. Risorse aggiuntive che non sono nella disponibilità delle istituzioni democratiche europee - leggi il Parlamento - ma solo degli Stati membri. Risorse indispensabili per l'avvio di una cooperazione strutturata permanente per rafforzare la sicurezza e la difesa europea, altro ambizioso obiettivo di questo Consiglio europeo, che recuperi lo spirito originario dell'Unione europea, che considerava la difesa comune come uno dei pilastri su cui costruire l'Europa unita e il cui fallimento pesa ancora come un macigno sull'integrazione politica dell'Europa. Su queste grandi questioni del nostro tempo si gioca il futuro dell'Unione, che non può non rispondere alla domanda su come proseguire nel cammino di integrazione. Come dal presidente Gentiloni Silveri già ricordato in altre occasioni e come ribadito dal presidente Tusk nei giorni scorsi in vista del prossimo Consiglio europeo, non si deve abbandonare l'obiettivo di portare i 27 su posizioni condivise, che rilancino il processo di integrazione. Tuttavia, da convinto sostenitore del sogno federalista, dico che non possiamo rimanere prigionieri dei nostri pur giusti principi, soprattutto quando l'alternativa è la paralisi, peggio ancora se è frutto di un modo distorto di concepire ed esercitare la propria appartenenza all'Unione. Contro chi blocca ogni ipotesi di riforma del diritto comune di asilo, di politica comune sui migranti, sul controllo e la sicurezza delle frontiere esterne, sul completamento del mercato unico, ivi compreso quello digitale, sull'istituzione di una *web tax* che ripristini le pari opportunità nel mercato ed eviti *dumping* fiscali, interni ed esterni, e anche sulle politiche commerciali e sulla *governance* economica occorre facilitare meccanismi di cooperazione rafforzata, per consentire a chi vuole di andare avanti nella solidarietà europea. Non si tratta di cedere a un pragmatismo apatico, disancorato dai valori di riferimento del modello europeo, ma di avere ben presente che l'opinione pubblica richiede interventi adeguati ai problemi del nostro tempo. Una concretezza guidata dai valori fondanti dell'Unione europea, senza la quale questo ideale rischia di essere travolto. Solo così si riuscirà a dare risposte sulla sicurezza, sull'immigrazione, sulla riforma dell'eurozona, sull'Europa sociale, che sono i prossimi appuntamenti dei prossimi Consigli. Ciò non significa rinunciare a traghettare tutti i 27 *partner* verso un altro tempo della storia. Non possiamo rinunciare ad esercitare appieno la vocazione politica dell'Europa, anche nei confronti dei processi disgregativi degli Stati-nazione formatisi nel XVIII e XIX secolo, di ricorrenti rivendicazioni autonomiste, che senza un'adeguata *governance*, che richiede un'Europa politica, rischiano di diventare dei processi di disgregazione che, se privi di orizzonte, sono destinati a essere travolti da nuovi autoritarismi o a produrre (vedi la storia dell'Irlanda, dell'Alto Adige e dei Paesi baschi) un nuovo terrorismo. È nell'equilibrio tra ostinazione nel perseguimento dell'unità e il rispetto delle oggettive diversità che occorre trovare la strada per rendere sempre più attuale e convincente il sogno sogno europeo che oggi è in crisi. Ma la politica non è la mera presa d'atto dell'esistente: è lo strumento per far diventare realtà la speranza, per far comprendere che si può. È l'esercizio paziente della ricerca degli strumenti migliori per raggiungere il fine, purché si abbia chiaro quale sia il fine che si persegue, e ciò negli ultimi anni non è sempre stato così chiaro. È con questo auspicio che ci auguriamo che il Parlamento possa accompagnare il suo sforzo, signor Presidente del Consiglio, e quello del Governo, che è stato oggi così presente in quest'Aula, con autorevolezza, e che vogliamo continui in questo suo sforzo per l'Europa unita e per una maggiore integrazione.

al Governo sono stati chiesti dei chiarimenti che vorrei brevemente fornire. Al senatore Monti vorrei ricordare nuovamente che il Governo ha preso posizione sul futuro bilancio dell'Unione europea con un *paper* presentato in aprile e ricordo anche che quando parliamo di riformare la zona euro non intendiamo semplicemente l'unione economica e monetaria, ma vogliamo rimettere in discussione anche alcune regole esistenti. Per questo abbiamo sollevato un dibattito sulle regole 2011 ed anche su vari aspetti del *fiscal compact.* Al senatore Paolo

quindi fino al 2023. È inutile lanciare cifre: sta ai britannici dirci quali sono i criteri per affrontare questo tema, che è fondamentale. Così come fondamentale è il tema

altri cittadini dell'Unione europea nel Regno Unito. Sono quindi pienamente d'accordo con il suo invito e, anche forti del vostro lavoro, proseguiamo nel negoziato, a livello tecnico, su questo aspetto. Ci sono dei passi avanti, come il riconoscimento riconoscimento da parte dei britannici del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea e dell'effetto diretto delle sentenze della Corte riguardanti i diritti dei nostri cittadini. Presidente, l'altro punto su cui credo di dover rispondere è

con il Comune di Milano e il sindaco Sala e con tutti i portatori di interesse del settore privato, sta facendo un lavoro di squadra molto intenso in una gara molto competitiva. Stiamo affrontando cercando di sfruttare al meglio la potenzialità di Milano, però purtroppo non è l'unica candidatura. Ce ne sono altre 19 e direi che sulle dita della mano o di una mano - senatore l'articolo, determinativo o indeterminativo - se ne contano altre con cui dobbiamo confrontarci. Certamente condivido con lei le valutazioni che ha fatto sulla forza della candidatura di Milano. infine, al senatore Santangelo. Ci sono dei punti specifici sulla difesa. Li ricordo anche per lasciarli agli atti: i *leader* discuteranno della creazione del Fondo europeo della difesa difesa e della proposta legislativa per un programma di sviluppo industriale della difesa europea. L'obiettivo, che credo si raggiungerà, è di adottare la proposta legislativa e di avviare anche il Fondo entro la fine dell'anno, dell'anno, anche alla luce delle conclusioni che potranno venire e che l'Italia auspica nel vertice di domani e venerdì, perché noi condividiamo in pieno

Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, credo che le risoluzioni riflettano la pochezza del dibattito odierno e soprattutto - lo devo dire con dispiacere - la pochezza delle comunicazioni venute dal Presidente del Consiglio. Sono stati toccati tre punti in maniera del tutto insoddisfacente. Dire che l'Italia è sempre stata un Paese che ha ricercato un maggior livello di integrazione è dire un'ovvietà che francamente non è degna di essere ascoltata in quest'Aula. Il problema è come arrivare a questo maggior livello di integrazione.

che poi De Gasperi, da una parte, e Altiero Spinelli, dall'altra, hanno declinato con alcune diversità. Questo schema è fallito, collega Susta, proprio sulla politica di difesa, ed è fallito proprio perché, in realtà, non si è risolto il problema della creazione di un nucleo di potere politico condiviso. In qualche modo, l'esercito europeo aveva lo stesso baco della moneta unica: sono stati fatti passi più lunghi senza che si risolvesse il problema del nucleo politico che doveva guidare e dare un indirizzo a questi passi. Dai Trattati di Roma in poi il problema dell'integrazione europea è stato risolto in un altro modo, cioè attraverso quello che viene chiamato il metodo Monnet: si trova un problema che in qualche modo viene compreso dalle popolazioni europee e si cede il livello di sovranità indispensabile per risolverlo, poi si parte da quel livello di cessione di sovranità per risolverne uno più complesso, in modo tale che la sovranità si può trasferire. Quello che è accaduto

da nessun altro nucleo di potere politico e per questo si è dispersa. Quello che ci aspettiamo quando si parla di trovare la strada per porci nella scia di quanto ha fatto il nostro Paese è che ci venga indicata una nuova ricetta. Come si crea questo maggiore livello d'integrazione, al di là degli *slogan* e dell'appello a un passato che non può più tornare, perché la situazione del mondo è cambiata e perché la situazione dell'Europa rispetto a quel mondo è cambiata?

sono un modello, sono principi che dovrebbero ispirare una politica. Questa politica non c'è, non ce l'ha il nostro Paese e non ce l'ha l'Europa. Francamente, sarà certamente non sufficiente, non commendevole una politica che propone soltanto di sigillare le frontiere, una politica che tende a difendere insieme i confini d'Europa non è stata ancora indicata e non mi sembra che abbiamo avuto alcun elemento in più

quasi vacuo questo intervento in dichiarazione di voto. Già, perché avremmo voluto interloquire con il Governo ma purtroppo abbiamo visto che, da ormai più di due ore, sia il Presidente del Consiglio dei ministri che tutti gli altri Ministri se ne sono andati, lasciando due Sottosegretari. Sottosegretari. È una questione di rispetto nei confronti delle tematiche e degli argomenti posti. Io vorrei parlare e vorrei che fosse riportata in Europa la voce delle imprese italiane che non riescono più ad operare sul mercato e non solo quelle grandi ma quelle più piccole, le piccole e medie imprese, come dico tutte le volte che ce n'è occasione in Commissione: da quelle agricole per passare a quelle industriali e a quelle artigiane. Io avrei voluto interloquire su questi aspetti con il Governo,

- ahimè - in un'Europa che voi, invece, declinate come la soluzione di tutti i problemi. Di queste cose avremmo voluto parlare con Ministri che qui non ci sono. Sottosegretario Gozi, dove sono i Ministri del suo Governo? Li abbiamo visti, certo, sul treno con Renzi.

chiuse), a destra e sinistra per fare propaganda elettorale insieme al segretario del partito, disertando la seduta del Senato dove ci si deve relazionare con il Parlamento per le priorità che il Governo deve portare in Europa per il nostro Paese. Non siete seri. Non siete seri, mancate di serietà! E capisco che arrivando alla fine di questa legislatura, ormai vi manchi anche il senso del ridicolo, - accidenti - in una circostanza come questa, lasciare tutti quei banchi deserti, che serietà dimostra nei confronti del Paese? Questa è la stessa serietà che vi porta oggi a dire che la priorità del vostro Governo è lo *ius soli*, non l'interesse dei cittadini italiani. Andate in Europa a dire che la vostra priorità e quello "0,0 e qualcosa" sul PIL

Ma come fate, nei confronti di un Paese che, invece, vi indica in tutti i modi le proprie priorità? Sottosegretario Gozi, in queste stesse ore, in questi giorni, abbiamo potuto vedere ancora una volta che cosa accade quando i nostri cittadini, non tutelati, si trovano a doversi difendere da soli.

Dopo lasciate i nostri concittadini a difendersi a mani nude o come possono, con un sistema che non li tutela neppure. Le priorità si chiamano legge sulla legittima difesa, abbassare il costo del lavoro, si chiamano diritti, diritti, gli stessi diritti di un lavoratore che, dopo aver lavorato tutta la vita, non ha la pensione e ha bisogno di andare a chiedere l'Ape social, dopodiché si trova respinta pure la domanda. Siete ridicoli! È su queste cose che dovete essere credibili quando vi confrontate in Europa. Il problema è che non avete la consapevolezza del ruolo che dovete rivestire nei confronti degli altri Paesi europei. I cittadini sono molto più maturi di voi. Vogliono democrazia, vogliono partecipazione e ve lo dimostreranno la prossima primavera, alle elezioni, quando vi cacceranno a casa, ma lo dimostrano già oggi, volendo partecipare democraticamente ad un *referendum* che si svolgerà in Lombardia e in Veneto, perché l'autonomia che si richiede in quelle Regioni non è nient'altro che la libertà di poter fare impresa, di poter avere le risorse per operare nell'economia, di poter coprire i costi sociali di cui oggi il Governo si dimentica, di poter dotare quelle realtà di infrastrutture di cui oggi il Governo si dimentica, nonostante ci siano tasse pagate per decine di miliardi di euro. non è nascondendo la spazzatura sotto il tappeto che si risolvono i problemi, non è negando il problema dell'incapacità del Governo nella gestione dei flussi di immigrazione clandestina che dimostrate serietà. Sottosegretario Gozi, nello schema di decreto legislativo che avete presentato oggi in Commissione per chiederne il parere, con cui rivisitate la composizione delle commissioni che devono valutare chi ha realmente diritto ad essere riconosciuto come profugo, che cosa fate? Aumentate le commissioni? No. Rivedete i componenti, togliete il poliziotto e il rappresentante delle amministrazioni locali per metterci due funzionari del Ministero dell'interno che possano, a comando, decidere e sveltire le pratiche. Questo è quello che voi fate e questo il vostro modo di essere seri. seri. Certo, le statistiche alla fine diranno che il sistema italiano funziona, andrete in Europa ed essa vi applaudirà, e gli italiani continueranno a pagare di loro tasca la vostra incapacità di decidere di governare. A casa dovete andare, altro che a Bruxelles!

nell'aeroporto di Mogadiscio ci sono più *jet* privati di quelli presenti negli *hangar* di Nizza. Ciò per dire che le ricchezze lì ci sono, ma sono distribuite in modo anomalo: tanti sono i poveri e pochissimi i ricchi. È per tale ragione che con la nostra risoluzione vogliamo che il Governo si impegni, anche a livello delle Nazioni Unite e dell'Unione europea per portare in quei

garantire, far capire e formare in Italia la consapevolezza che con i meriti e i bisogni si può andare avanti e progredire.

l'apprezzamento del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE per le parole del Presidente del Consiglio e il sostegno all'azione del Governo in sede europea. Mi limito a ribadire che è importante che l'Europa metta al centro la ripresa economica, il sostegno all'Italia nella gestione della crisi migratoria, perché troppo spesso siamo stati lasciati soli. Abbiamo apprezzato il lavoro efficace svolto in questi mesi, ma oggi il nostro Paese ha bisogno dell'aiuto dei *partner* europei. Sulla politica economica dobbiamo spingere con ancora maggiore convinzione su tutte le misure che aumentino la crescita. I dati, per quanto positivi, non sono ancora in grado di attutire il colpo inferto al nostro sistema negli anni Infine, sulla questione catalana, rinnovo l'invito espresso anche dal presidente Zeller ad un maggior interventismo italiano ed europeo. Si lavori affinché si riapra un confronto tra Madrid e Barcellona, riconoscendo le istanze di autogoverno del popolo catalano e scongiurando una crisi, i cui effetti, per tutta l'Europa, potrebbero essere imprevedibili, con un vero e proprio effetto domino. Allo stesso tempo è importante che l'Europa giochi il suo ruolo nel mondo, come elemento di stabilizzazione rispetto alle grandi tensioni, dalla Corea, all'Iran, ma anche nel rapporto con la Turchia.

regolamento di Dublino e la posizione della Turchia in questa vicenda, sia per quanto riguarda la *web tax*, perché anche noi chiediamo che si arrivi ad una definizione condivisa di iniziative di tassazione dei cosiddetti *over the top*, ovvero dei grandi operatori, sulle piattaforme Internet europee, da un punto di vista economico.

alla necessità di ribadire un secco diniego a qualsiasi ipotesi, al momento, di adesione della Turchia all'Unione europea, dato quello che sta avvenendo in quel Paese in termini di tutela e di garanzia dei diritti dei cittadini. Siamo d'accordo anche sulla necessità di dare esecuzione effettiva ai rimpatri per coloro ai quali non è stato riconosciuto il diritto di protezione internazionale, e come pure sulla necessità di invocare, in ambito europeo, l'adozione di politiche che scoraggino iniziative fortemente lesive nei confronti delle minoranze linguistiche e quindi anche i relativi conflitti. Non siamo

né quello relativo ad a una nostra eventuale adesione all'Eurocorpo e quindi a far parte di un embrione di esercito comune. Non siamo d'accordo sulla promozione, in questo momento, di una riflessione sul ruolo della Turchia che possa andare nella direzione di una sua adesione alla Comunità europea. Siamo molto scettici anche sulla fumosità con cui hanno elaborato altri impegni nei confronti del Governo, come quelli che riguardano la gestione dei flussi migratori e la

il sostegno della candidatura di Milano come futura sede dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA). Quindi, ci asterremo

che vada in direzione della ricerca, perché sappiamo che quando parliamo di Brexit uno degli aspetti molto importanti che riguarderà la trattativa è proprio quello della ricerca universitaria e scientifica. Sappiamo che il Regno Unito, e in particolare la Gran Bretagna, percepiscono molti molti finanziamenti dall'Unione europea in tal senso, perché i loro atenei sono tra i più appetibili in Europa e quindi c'è molta preoccupazione nel mondo della ricerca sulla libera circolazione dei ricercatori e sui progetti che sono nati e stanno andando avanti in cooperazione tra atenei europei - quindi non solo italiani

che il ruolo delle ONG è stato ambiguo e di favoreggiamento sostanziale alle attività degli scafisti. Poi c'è stato il famoso regolamento che abbiamo votato all'unanimità - atto eccezionale nella storia di questa legislatura - in Commissione difesa, e discusso anche in Aula, che è stato alla base delle azioni del Governo che hanno portato a una riduzione sensibile degli sbarchi, che in questi ultimi giorni invece stanno riprendendo a causa della confusione che si è creata e della situazione che riguarda la Tunisia. proposta di risoluzione, che noi ovviamente voteremo, insieme a quella del Gruppo della Lega Nord (le altre non le voteremo), richiama anche, sottosegretario Gozi, a una serie di doveri: ad esempio, la questione delle sanzioni nei confronti della Russia, ossia una scelta che sta danneggiando l'Italia e

importantissimo, e questo dovrebbe spingere ancora di più a riprendere dei pieni rapporti. Nella nostra proposta di risoluzione abbiamo richiamato il rischio dell'arrivo dei *foreign fighter*, la necessità di una voce unica europea, e non ripeto le cose molto chiare dette oggi dal presidente Romani circa il ruolo ambiguo di altri Paesi europei e la debolezza italiana nell'esigere una convergenza sui nostri sforzi. Per quanto riguarda altri temi, vogliamo che si passi veramente a decisioni concrete sulla *web tax*. C'è una impunità fiscale per alcune realtà dei giganti della rete, i cosiddetti che oramai è intollerabile e che è stata evidente anche in questi ultimi mesi, creando una sperequazione rispetto a situazioni di pressioni fiscali intollerabili su artigiani e su attività di commercio. Vogliamo inoltre rivendicare nei confronti dei rappresentanti del Governo il ruolo decisivo, non che la nostra parte politica ma che le istituzioni europee stanno svolgendo su alcuni temi delicati: penso alla vicenda degli NPL (che oggi hanno un altro nome), delle sofferenze bancarie. L'azione ingiusta, sbagliata, vessatoria nei confronti delle nostre banche che alcuni esponenti di seconda fila

quando dalla BCE sono state prese decisioni che, se venissero applicate, strozzerebbero le nostre imprese, la possibilità di erogare credito? Vogliamo pertanto rivendicare la nostra azione e la nostra posizione, posizione, e sperare che il Governo italiano sostenga l'azione che nel Parlamento europeo ha assunto, nel suo ruolo istituzionale e non di parte, il presidente Tajani; iniziative sulle quali vediamo il Governo molto esitante e balbettante.

questa opportunità, che sarebbe di grande importanza non solo sotto il profilo del segnale morale, ma anche del significato economico, della ricerca che questa localizzazione avrebbe nella città di Milano. Infine, oggi noi abbiamo richiamato anche il tema dello *ius soli* e della cittadinanza. Non ripeto quanto è stato detto, ma noi ci auguriamo che si eviti quella che è una scelta sbagliata anche nel contesto europeo. europeo. Il tema della cittadinanza, infatti, come si fa a non discuterlo a livello europeo? Che senso ha una fuga in avanti italiana con una eventuale legge demagogica, quando siamo nel tempo di Schengen e nel tempo della libera circolazione?

guidati da Berlusconi. Poi altri Paesi europei o gli americani vollero guerre sbagliate e le cose sono andate come sono andate. Sulla cittadinanza bisogna discutere, sì, ma a livello europeo perché una fuga in avanti italiana sarebbe sciagurata. Noi vi invitiamo a non farlo: non solo perché, probabilmente, non avete i numeri in quest'Aula, ma perché non li avete neanche nel Paese, dove una scelta demagogica di quel tipo diventerebbe la ragione di un grande *referendum* abrogativo e sarebbe il principale il principale argomento della campagna elettorale. Quindi, noi abbiamo una duplice possibilità di vittoria: vincere la battaglia politica, evitando leggi italiane ma con una riflessione europea, che si connette ai temi che stiamo discutendo oggi; se volete andare avanti a colpi di fiducia, sarebbe il Paese a darvi la risposta nelle urne delle elezioni e nelle iniziative democratiche per abrogare leggi sbagliate.

perché esse hanno l'obiettivo di sostenere e rafforzare la complessiva azione dell'Esecutivo sulla scena europea ed internazionale anche in occasione di questo Consiglio europeo. Sui temi disparati, rilevanti e cruciali che saranno all'ordine del giorno domani e dopodomani sono stati raggiunti negli ultimi tempi dei primi significativi risultati, grazie anche alla forte e costante iniziativa italiana. Si tratta oggi di insistere, di non mollare la presa e di spingere ancora più avanti la situazione e la realizzazione. Sulle migrazioni occorre continuare con impegno per qualificare il ruolo dell'Europa senza lasciare soli

Si tratta di stanziare più risorse per l'integrazione dei migranti accolti in Europa, anche attraverso il rifinanziamento del *trust fund* dell'Unione europea e gli accordi con i Paesi africani. Sul digitale occorre proseguire sulle priorità definite a Tallinn, in particolare sulla creazione di piattaforme europee per le piccole e medie imprese perché sia presentata al più presto una proposta condivisa sulla *web tax*, sulla quale vi è il totale consenso del nostro Gruppo. Sulla questione della difesa occorre dare seguito al progetto PESCO, per non disperdere il patrimonio industriale nel settore della difesa del nostro Paese e per sostenere la richiesta che l'Italia diventi membro effettivo dell'Eurocorpo, visto che siamo il Paese più esposto verso l'Africa ed il Medio Oriente, e per realizzare concretamente una procura antiterrorismo europea. Sono tutti obiettivi importanti. Infine, è giusto, come ha detto il presidente Gentiloni Silveri, continuare ad avere rapporti costruttivi con il Regno Unito, ma occorre grande fermezza sugli obiettivi della transizione, in particolare per i nostri cittadini. Tutti questi impegni richiamano l'esigenza di un'azione più forte, coordinata e unitaria dell'Europa. Non ci sarà azione efficace su migrazione, digitale, difesa o altro senza una visione comune e un impegno corale, senza istituzioni, politiche e strumenti sempre più comunitari e meno frammentati. L'Italia ha un ruolo forte da giocare perché è un Paese fondatore, ha il prestigio e la responsabilità e perché è anche nel suo precipuo interesse. Dobbiamo farlo in un momento assai delicato, ma anche portatore di nuove opportunità. Ci sono speranze e criticità. Le speranze sono quelle di una ripresa meno effimera forse di quello che pensavamo, che dia impulso all'occupazione e alla coesione sociale, le speranze sono anche quelle di nuovi impegni, segnati in particolare negli ultimi tempi dagli interventi di Juncker e Macron, che dimostrano che comincia a esserci un dibattito europeista di spessore più alto, a cui anche noi partecipiamo e dobbiamo continuare a partecipare. Ci sono anche le criticità e le tensioni, se mettiamo insieme le vicende della Catalogna (per la quale auspichiamo un dialogo costruttivo, che salvi l'unità del Paese e rafforzi l'autonomia della Catalogna stessa, evitando di innescare un processo disgregativo che sarebbe negativo per l'Europa), le elezioni in Germania e in Austria, che vedono crescere le forze antieuropee e le asperità del negoziato sulla Brexit, di cui ha parlato in Senato il capo negoziatore per l'Europa Michel Barnier. Queste difficoltà dicono della distanza che ancora separa l'Europa, la sua immagine e la sua iniziativa dal sentimento popolare. Ma è proprio in questi passaggi critici che dobbiamo saper rilanciare e guardare più avanti.

desidero concludere dicendo che è giusto e necessario criticare l'Europa per le sue debolezze e manchevolezze, nonché per la sua burocrazia e i suoi egoismi, ma è ancora più giusto, necessario e urgente lavorare per ricostruire e farsi parte attiva affinché i processi di consolidamento e rinnovamento dell'Unione vadano avanti. Essere come Italia soggetto attivo aiuta l'Europa e contrasta i rischi dell'*empasse* e del ripiegamento - e questo è già un patrimonio importante per tutti noi e, peraltro, rafforza il nostro ruolo di soggetto che crede nell'Europa e la vuole fermamente, sia pure su basi più democratiche, efficaci e strategiche. L'impegno del Governo sui temi del Consiglio europeo e sul rilancio dell'Europa servono all'Italia e a tutti noi. Fuori da questo quadro non troveremo le risposte ai nostri problemi.

risultata vincitrice del bando per l'assegnazione di quel posto di insegnamento. Allora è chiaro che una delle concorrenti, la dottoressa Alessandra Castellani, ha fatto ricorso contro il risultato di questa graduatoria, poiché è palese che qualcosa non andava. Non è possibile è possibile che chi presiede la commissione valutatrice sia poi anche la stessa alla quale viene assegnato l'incarico di insegnamento; c'è un lievissimo conflitto di interessi.

un fiore all'occhiello per Faenza, per l'Emilia-Romagna e anche per l'Italia intera, in teoria, perché lì si sono formati grandi artisti artisti e grandi ceramisti. Sappiamo, però, che questo comparto verte ormai da anni nell'anarchia più totale; al suo interno vi sono non solo conflitti di interessi, ma anche sperperi di denari pubblici dovuti, ad esempio, all'attivazione di corsi inutili; inutili; ci sono conflitti di interesse legati, ad esempio, alla somministrazione di corsi di italiano per studenti cinesi; ci sono problemi nello smaltimento delle delle sostanze che vengono utilizzate nei laboratori di incisione, che sono particolari e dovrebbero essere smaltite in sedi apposite, con pratiche adeguate;

delle belle arti e in tutte le istituzioni di alta formazione; scoprirà delle belle cose, scoprirà quanto avevamo ragione noi.

Questo è quello che è successo il giorno 11 ottobre 2013, quando un barcone carico di uomini, donne e bambini in fuga da una guerra oscena in Siria si è rovesciato a Sud di Lampedusa. Circa 60 di loro erano pericolosissimi bambini. E questo paragone, se non altro, ci impedirà, vi impedirà di girare la testa dall'altra parte. Il dolore dei familiari deve essere lenito. Numerose prove accusano alti ufficiali della Marina e, poiché ogni dubbio deve essere sollevato dalla istituzione Marina militare, ho depositato una interrogazione ai vari Ministeri, dopo le ulteriori e decisive prove emerse. Un'interrogazione dettagliata con cui si chiede cosa intenda fare la ministra Pinotti per fugare ogni ombra di dubbio. Le chiediamo di attivarsi per ottenere i documenti e le registrazioni custoditi dalle autorità maltesi e dalla nave Libra, nave quel giorno più volte chiamata via radio sul canale 16 di soccorso marittimo dal velivolo militare delle forze armate maltesi. Eppure, il pilota ha dichiarato che vedeva sia la nave Libra che il barcone, poiché erano vicine, ma che la nave militare italiana non rispondeva. La Libra arriverà solo alle ore 18, poiché da Roma, come dimostrano le registrazioni, le era stato addirittura ordinato di allontanarsi dalla scena. Chiediamo alla ministra Pinotti cosa intenda fare nei confronti di chi le fece riferire il falso in Aula il 17 maggio 2017, visto che già erano di dominio pubblico tutte le comunicazioni, le foto e i filmati che documentano quella tragedia. Cosa intenda fare riguardo al capo di stato maggiore della Marina militare, ammiraglio Girardelli, che due giorni fa ha dichiarato: «siamo sereni (...) sicuri di aver fatto comunque il nostro dovere». Le chiediamo, soprattutto, di evitare dì prendere in giro l'intelligenza degli italiani, rifugiandosi dietro la risibile scusa che il mancato salvataggio del barcone sia dovuto a discussioni burocratiche, come ha detto l'altro ieri. Scusa risibile, poiché non vi fu alcun contrasto, opposizione o dialettica tra italiani e maltesi, come dimostrano le registrazioni. Il fatto è semplice: ci fu una richiesta di soccorso dal barcone, attraverso il dottor Jammo, che alle ore 12,39 comunicò chiaramente la situazione di pericolo imminente in cui si trovavano, comunicò le coordinate e che a bordo vi erano bambini feriti e disse che stavano affondando. La situazione era chiara da subito. Come Come risultato abbiamo che la nave più vicina, la nave Libra della Marina militare che avrebbe potuto salvare tutti in trenta, quaranta minuti, lascia che il barcone si rovesci ed arriva sulla scena del disastro alle ore 18, quando oramai 268 persone erano morte. Ricordo: 60 bambini, signor Presidente, 60 bambini. Dobbiamo dire altro? Presidente, sabato scorso, in anteprima ho visto il film documentario «Un unico destino», che il giornalista Fabrizio Gatti ha realizzato dopo quattro anni di indagini. È un documento chiaro e agghiacciante. Il ghiaccio che mi ha scosso le vene quella sera sia lo stesso di chi deve agire nel nome della giustizia e della verità. giustizia e della verità. Affinché questa tragedia non sia archiviata - e il rischio è altissimo - ognuno deve corrispondere con dignità ed onore alle responsabilità del proprio ruolo. Si difendano le istituzioni, Presidente, non le persone. *(Applausi